delle Commissioni riunite che si sono conclusi alle ore 5,30 di questa mattina e come già comunicato ai Gruppi, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12 con le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori e la discussione del decreto-legge semplificazioni. La seduta è sospesa. *(La seduta, sospesa

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 10 settembre. Resta confermato, per questa settimana, l'esame fino alla sua conclusione

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede, alle ore 16, le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi tre ore, incluse le dichiarazioni di voto. Il calendario della prossima settimana prevede, a partire da martedì 8 settembre, la discussione dei seguenti argomenti: relazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio sulla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio; ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri; prima deliberazione sul disegno di legge costituzionale concernente l'estensione dell'elettorato per il Senato, già approvato dalla Camera dei deputati; sindacato ispettivo. Giovedì 10 settembre, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Una seconda questione riguarda

proponiamo che il voto di fiducia si svolga non venerdì, ma quando il Governo sarà pronto, e cioè - speriamo - lunedì. In ogni caso, i lavori della Camera saranno evidentemente più che compressi, ma è chiaro che onorevoli senatori e senatrici, la proposta della Lega sul calendario anzitutto - così com'era stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo prima della pausa estiva - che il presidente del Consiglio Conte venga in Aula a riferire sul contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

che la fiducia non venga votata venerdì mattina - siamo anche noi convinti che il maxiemendamento non sarà pronto per le ore 9,30 di venerdì, così come calendarizzato

assolutamente ingiustificato che, dopo tutto quello che è venuto fuori dai verbali del Comitato tecnico-scientifico,

C'è un verbale che ha circa 3.400 o 3.500 allegati. Vogliamo tutti gli allegati e, quindi, che Conte venga in Assemblea a rispondere del perché non ha ancora desecretato gli atti.

sul tavolo del Governo giaceva uno studio della Fondazione Bruno Kessler, che sostanzialmente prevedeva, in modo azzeccato, tutto quello che sarebbe successo e addirittura anche

e pochi giorni dopo questo materiale risulterà essere introvabile. Queste sono risposte che il Presidente del Consiglio deve venire a dare in Parlamento, se davvero è una persona seria, come crede di essere o come si dipinge.

con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si autorizzi la Tim a utilizzare i dati sensibili del 5G, attraverso la tecnologia cinese Huawei, mettendo a rischio e a repentaglio la sicurezza nazionale, senza

quante persone sono state contagiate in discoteca, quante persone sono state contagiate tra gli immigrati. Vogliamo sapere quanti sono in terapia intensiva. Vogliamo dati chiari e certi, perché la popolazione italiana vuole trasparenza e chiarezza nelle idee che vengono portate avanti!

Ci sono le scorte per i vaccini antinfluenzali? Ci sono le scorte di farmaci? Ci sono le scorte di mascherine? Ci sono le scorte di bombole d'ossigeno? Abbiamo i *triage* pronti, fuori da tutti gli ospedali, per accogliere eventuali pazienti Covid, senza che debbano entrare al pronto soccorso? Abbiamo impostato una campagna informativa? Siamo pronti, sì o no? No, perché il piano non c'è, altrimenti sareste già venuti in Aula a portarcelo. Ma venite almeno a spiegare perché, dopo sei mesi, non avete ancora un piano chiaro che faccia in modo tale

non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare; dobbiamo essere duri e inflessibili; non si entra in Italia in quel modo e, soprattutto in questo momento di fase acuta,

si perdono le tracce; e soprattutto ci spieghi come sia possibile che in un *hotspot* di 192 posti vengano assembrati e schiacciati 1.500 immigrati. *(Applausi)*. Questo è uno scandalo, a testimonianza che l'ideologia

o razzismo e quant'altro! *(Applausi)*. Qui l'importante è mettersi la coscienza a posto, che è anche un po' di moda e un po' *radical chic*; poi, una volta che sono sbarcati, che facciano la fine che devono fare e non ci interessa nulla. Vergogna! Conte, vieni in Aula! Ti devi vergognare! Vieni a rispondere alle domande che il popolo italiano ti sta ponendo! *(Applausi)*.

tornata da Malta, non stando bene, viene ricoverata, si aggrava e finisce in terapia intensiva. Si trattava di una *fake news* di quelle clamorose,

c'era. Io ho chiamato l'ospedale Cervello e ho chiesto quanti pazienti sono in terapia intensiva: la direzione sanitaria mi ha detto «zero». Era una *fake news*, come le altre che ho appena citato.

Alla Gavi Foundation di Bill Gates credo abbiate dato dai 180 ai 400 milioni, mentre al professor De Donno avete inviato i NAS.

nel mondo ci sono 11 milioni di morti l'anno tra tabacco e alcol, c'è un disegno di legge interessante.

998 reca: «Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata tramite la legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati»,

Scusi, lei adesso si sieda e permetta agli altri di parlare. Ha già parlato. Non capisco la polemica fuori microfono. Signor Presidente, colleghi, Governo, la Conferenza dei Capigruppo svoltasi ieri ha sciolto molti nodi importanti, ma - come si è già potuto percepire dagli interventi che mi hanno preceduto - quella di oggi non è soltanto una discussione sul calendario; non è soltanto la discussione - sia pure importante e ci arriverò

ad ogni evidenza una discussione di carattere politico. Prima di affrontare il nodo politico che riguarda la giornata di oggi, voglio immediatamente dire quali sono le proposte di modifica di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il calendario. E poi le sosterrò con un ragionamento politico che appunto nasce e riguarda la giornata di oggi. Fratelli d'Italia chiede che il presidente Conte venga in Aula per delle comunicazioni - come già previsto prima della sospensione estiva dell'attività del Parlamento - a rispondere all'Assemblea

come quella in cui richiedere il voto di fiducia; poi si è slittati a venerdì. C'è una considerazione da fare: troppe volte siamo stati in quest'Aula

molto più saggio e opportuno indicare con precisione i termini di presentazione della richiesta del voto di fiducia e la sua celebrazione,

spostare il voto di fiducia indicato per venerdì. Vengo all'ultima richiesta e poi entrerò nel merito. Fratelli d'Italia per la settimana prossima ha già richiesto che venga calendarizzato

derubricato e modificato, indicando nella figura del ministro Speranza colui che è stato designato a tenere le comunicazioni in Assemblea. Sostanzialmente il presidente Conte non verrà,

quando, per quanto tempo (chiudendo per i seggi elettorali), su quali autobus, con quanti congiunti improvvisati, quante ore faranno, dove mangeranno, se andranno in palestra? palestra? Vi rendete conto che dietro ogni alunno ci sono famiglie, ci sono genitori che devono tornare al lavoro, ci sono *baby-sitter* da contrattualizzare? Vi rendete conto che ci sono ragazzi che devono iniziare i primi cicli del liceo e delle medie, in prima elementare? Stiamo mandando in prima elementare dei bambini che sono stati a casa mesi e non sono stati prescolarizzati. Vogliamo considerare l'ingresso in prima elementare come un momento delicato? Rispetto a queste domande di comune buon senso, quali sono le risposte? L'inizio della scuola ha preso il Governo alla sprovvista come se fosse una calamità naturale. L'inizio della scuola era un fatto prevedibile e previsto rispetto al quale il Governo si è dimostrato totalmente inadeguato. Ci avete detto che avreste trovato sedi per i seggi elettorali; poi ci avete detto che non le avete trovate; ci avete parlato di banchi di legno da dividere in due, e poi sono arrivati quelli con le rotelle. Abbiamo messo l'Esercito a scaricare i banchi delle scuole come se fosse un'emergenza naturale. *(Applausi)*. Ma quale emergenza? La scuola cominciava: lo dovevate sapere e vi dovevate organizzare. E allora scuole,

domande che aspettano una risposta perché dalle relative decisioni, dalle decisioni che il Governo non prende e non comunica, dipende la vita quotidiana delle persone.

la sua assenza una fuga, anche perché non è una questione di impegni. Questa assenza si contestualizza con tutto il resto; si contestualizza con quanto è accaduto ieri alla Camera, con la dittatura sanitaria con la quale si prolungano i termini dell'emergenza; si contestualizza con la richiesta continua di voti di fiducia: ieri sul

per cento dei testi in possesso della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativi a tutto quanto ha riguardato l'emergenza Covid e al suo passaggio dall'epidemia alla pandemia. Bisogna fare chiarezza. I cittadini italiani hanno diritto di sapere e bisogna cominciare a rispondere in Aula e non nascondersi. L'assenza

adesso siamo alla fuga rispetto alle responsabilità, davanti a un Paese in ginocchio dal punto di vista economico per la pandemia e lungamente provato. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia

a loro dire, è chiamato a rispondere a molte questioni rimaste irrisolte, non solo relative alla pandemia. Si riferiscono all'utilizzo del MES, alla desecretazione dei verbali e degli allegati del Comitato tecnico-scientifico, alle questioni degli immigrati e della scuola. inoltre, che il voto finale sul decreto semplificazioni sia spostato da venerdì a lunedì prossimo.

Presidente, ci apprestiamo in una contingenza particolare a esaminare in Aula un provvedimento importante. Se già in circostanze diverse trattare della conversione di un decreto che riguarda i temi più disparati, tutti rilevanti e soprattutto destinati a incidere in maniera significativa sulla vita e l'agire quotidiano di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche richiederebbe attenzione e partecipazione, ciò diventa ancora più indispensabile nel delicato momento che il Paese sta attraversando. infatti con questo spirito che, prima di addentrarmi su considerazioni di merito, voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe, i rappresentanti del Governo, la Presidenza del Senato, i presidenti di Commissione Coltorti e Parrini e tutti gli Uffici del Senato e dei Gruppi parlamentari che, con la consueta competenza e dedizione, ci hanno assistiti per aver svolto, nel pieno della stagione estiva, un attento lavoro di esame, di verifica e miglioramento del testo che oggi ci apprestiamo a discutere in Aula dopo un articolato dibattito nelle Commissioni. *(Brusio)*. Presidente, così non riesco Senatrice, prosegua. Chi non è interessato a sentire la relazione può uscire dall'Aula in modo da non disturbare la relatrice. Il decreto-legge che stiamo esaminando, infatti, pur arrivando in una fase che - non c'è bisogno di dirlo - è ancora pesantemente contrassegnata dall'emergenza sanitaria e dalle sue pesanti ricadute sociali ed economiche, segna una nuova fase della risposta che le istituzioni sono chiamate a dare alla pandemia in termini legislativi. Per mutuare un'espressione impiegata in altro senso e contesto, inizia la fase 2, e cioè siamo al passaggio dalla fase della doverosa risposta all'emergenza a quella della ripartenza, al momento cioè in cui siamo chiamati ad offrire al Paese gli strumenti per tornare a guardare al futuro con ottimismo. Lo spirito della semplificazione è quello che ha ispirato il Governo nel formalizzare il decreto-legge. *(Brusio)*. Presidente, mi gridano dietro all'orecchio e non riesco a parlare. Per cortesia, si sta svolgendo la relazione sul decreto semplificazioni. Chi non è interessato - lo ripeto - può uscire tranquillamente dall'Aula, lasciando alla relatrice la possibilità d'intervenire. Diversamente non si capisce nulla.

Lo spirito della semplificazione è quello che ha ispirato il Governo nel formalizzare il decreto-legge ed è questo anche lo spirito - ne do atto alle colleghe e ai colleghi di tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione - che ha accompagnato il lavoro nelle Commissioni. Degli effetti sociali ed economici della pandemia si è detto molto e a volte anche a sproposito, ma non possiamo negare come in Italia la crisi che ne è seguita abbia messo ancora più in evidenza la fragilità e la criticità che affligge il nostro sistema economico, il rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini, la capacità competitiva delle imprese e quella complessiva del Paese. Siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno di un vero e forte cambio di prospettiva; uno scossone per rilanciare l'economia, liberare le energie produttive dalla tenaglia di una burocrazia farraginosa e sbloccare quelle infrastrutture di cui tutti abbiamo bisogno per tornare a crescere, per migliorare la qualità della vita e della competitività del nostro Paese. Paese. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare va in questa direzione: rompere il groviglio di procedure inutili, di veti, di norme ormai inapplicabili o comunque irragionevoli che hanno rappresentato un costante freno al potenziale di crescita del Paese e che, in un momento come quello attuale, rischiano di rappresentare un'inaccettabile zavorra, un ostacolo alla ripresa economica e occupazionale. Non è, né può essere ovviamente un punto d' arrivo, ma rappresenta certamente un forte, significativo e chiaro punto di partenza. Ed è proprio guardando alle tematiche fondamentali del provvedimento che si coglie il senso della direzione di marcia che ci si impone. Non è un caso, infatti, che la prima parte del testo, i primi dieci articoli, sia dedicata alla modifica e alla semplificazione delle procedure relative agli investimenti pubblici, intervenendo sulle criticità che ognuno di noi ha potuto riscontrare un po' a tutti i livelli sul territorio. procedure già di per sé spesso inutilmente complicate e suscettibili di incertezze interpretative, che alimentano un ricorso spropositato, quanto spesso temerario, alla giurisdizione. Tale generale rigidità di sistema, lungi dal tutelare l'interesse pubblico e la legalità, si risolve a solo svantaggio del territorio, dei cittadini e delle imprese. Si è perciò inteso agire su due fronti: da un lato, prevedendo misure mirate, volte allo sblocco della miriade di opere cantierabili e, in qualche caso, perfino avviate e rimaste ingiustificatamente incagliate, con procedure speciali, come prevedono gli articoli 8 dall'altro, introducendo a regime un diverso approccio che, fermo restando il rigoroso rispetto della legalità e della trasparenza, responsabilizzi le pubbliche amministrazioni, a iniziare dai dirigenti, quanto al completamento dei procedimenti. In altri termini, si propone di guardare alle infrastrutture non come fascicoli problematici, ma come risposta a esigenze inderogabili del nostro Paese. È in questo senso che si è voluto affrontare anche il punto dolente dei contenziosi in sede giurisdizionale e dei purtroppo frequentissimi casi di opere che restano sospese per tempi inaccettabilmente lunghi. Se alla giustizia amministrativa spetta valutare la legittimità delle procedure, è proprio a noi, come legislatori, che spetta di approntare un apparato normativo che garantisca il più importante degli interessi legittimi, quello generale dei cittadini a vedere le infrastrutture completate e fruibili e che il gettito delle proprie tasse non finisca sprecato in una delle troppe opere incompiute sparse nel nostro Paese.

La centralità dell'investire, del realizzare e del poter contare su tempi certi e procedure trasparenti si pone ugualmente per il settore privato. È questo lo spirito dell'articolo 10, che guarda all'attività edilizia in una prospettiva dinamica, in cui le esigenze di conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale non sono affatto sacrificate, ma sono invece esaltate guardando alla valorizzazione e alla riqualificazione e rigenerazione del tessuto edilizio esistente, come un corpo vivo e non come qualcosa da mandare in rovina, per poi magari indulgere follemente in un inaccettabile nuovo consumo di suolo. Quella stessa prospettiva dinamica e positiva si ritrova in tutta la parte relativa alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in cui istituti e strumenti già esistenti (dal silenzio-assenso ai termini procedimentali) vengono opportunatamente valorizzati e riportati pienamente alla loro funzione di garanzia del cittadino e dell'interesse pubblico, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa. È anche perseguendo questa prospettiva che l'introduzione di norme che finalmente disincentivano l'irrazionale proliferazione di oneri regolatori, unita a una decisa opzione per il *digital first*, rappresenta un passo in avanti per un diverso rapporto fra cittadini e imprese, da una parte, e pubblica amministrazione, dall'altra, dall'altra, che dev'essere basato sulla certezza delle regole e sulla semplicità delle procedure, a iniziare anche dalla stessa modulistica. Per ragioni di celerità non mi addentrerò nelle tante rilevanti previsioni in altre materie, come: università; trattamento economico degli appartenenti

erariale e penale dei pubblici funzionari. L'incertezza interpretativa, infatti, lungi dal tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, è stata fonte di confusione, di paura, a volte immotivata, di generale irresponsabilità e di un atteggiamento volto a procrastinare, quando non omettere, la doverosa azione. A ben guardare il rovescio della stessa medaglia, ai cittadini e alle imprese l'amministrazione deve riconoscere più fiducia e, viceversa, dev'essere pronta a controllare e intervenire concretamente in caso di abusi e distorsioni, non limitandosi a ostacolare l'iniziativa privata, per poi rimanere inerte in caso d'irregolarità. Ritengo importanti anche le innovazioni introdotte nella disciplina d'impresa con riferimento sia alle misure incentivanti sia a quelle destinate, fra l'altro, a facilitare la capitalizzazione. misura è giustificata dalla contingenza, ma si pone altresì in linea con l'obiettivo di rafforzare e modernizzare il nostro tessuto imprenditoriale, costituito soprattutto da piccole e medie imprese, nell'ottica di una competitività di più lungo periodo. Consentitemi poi di rivendicare come importante l'intervento sulle Zone economiche speciali (ZES) e la possibilità d'istituire Zone franche doganali (ZFD), strumento di vero stimolo alla crescita, in particolare per le zone insulari e costiere, che va di pari passo con le innovazioni introdotte nella disciplina portuale. In ultimo, ma non certo per importanza, c'è la parte dedicata all'ambiente, anche questa concepita in un'ottica integrata e di lungo dalla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale agli interventi per la diffusione e il consolidamento di un sistema energetico sostenibile, alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico. misure diverse e puntuali, spesso finalizzate anche ad armonizzare la normativa nazionale con l'evoluzione di quella comunitaria, ma accomunate dalla stessa prospettiva di cui ho detto prima: non una tutela basata solo e soprattutto su divieti, ma una valorizzazione attiva, tale per cui uno sviluppo sempre più pienamente sostenibile è il percorso obbligato per ritornare a crescere e la strada su cui indirizzare la ripresa economica dopo il duro colpo di questi mesi. mesi. È con questo spirito che, avviandomi a concludere, auspico che quest'Assemblea voglia esaminare e approvare il disegno di legge di conversione, che ha già raccolto - lo ribadisco - l'utilissimo contributo degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dai colleghi di tutti i Gruppi parlamentari e che arriva al nostro esame arricchito e migliorato. Proprio con riferimento ad alcune proposte emendative che non hanno potuto trovare accoglimento, anche per il carattere ordinamentale e non finanziario del decreto, il mio auspicio è che, assieme ad altre, possano essere indirizzate e valorizzate nei provvedimenti che ci troveremo ad esaminare in un prossimo futuro. futuro. Mi perdonerete se concludo ripetendomi: questo provvedimento è un passo importante, ma non conclusivo; è l'inizio di un cammino che, nel rispetto della diversità di ruoli e posizioni, ma nella comunanza di intenti, deve vederci lavorare al meglio delle nostre forze per rispondere a un Paese che guarda a noi,

Signor Presidente, prima di iniziare voglio ringraziare tutti i colleghi della 1a e dell'8a Commissione per il lavoro svolto in queste settimane, per l'ascolto e il recepimento dei suggerimenti pervenutici dagli auditi, dalle associazioni, dalle imprese, dal mondo dell'università e dalla pubblica amministrazione, al fine di dare concretezza e rendere davvero innovativo il testo in oggetto. Onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a discutere in quest'Aula, com'è desumibile dal titolo, nasce dall'esigenza di rendere questo Paese più semplice e veloce, sburocratizzando la farraginosa macchina amministrativa, rendendo più agevoli le procedure e dando supporto alla rivoluzione digitale della pubblica amministrazione. Questi obiettivi, già importanti considerando la situazione burocratica del nostro Paese, assumono maggiore valore perché hanno lo scopo di rendere maggiormente efficaci alcuni provvedimenti adottati per favorire la ripresa e dare nuovo impulso all'economia, puntando su settori chiave come l'edilizia e la *green economy*. Passando all'esame del testo, il nucleo centrale del provvedimento è costituito dalla semplificazione burocratica e dallo snellimento delle procedure amministrative, puntando su quattro cardini che corrispondono ai titoli in cui il decreto-legge è diviso: semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno alla diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazione in materia di attività d'impresa, ambiente e *green economy*. Si parte da un presupposto semplice: senza digitalizzazione non può esserci semplificazione. Per eliminare l'eccessivo carico burocratico in capo alle diramazioni pubbliche, il decreto-legge prevede nuove regole per favorire l'identità e il domicilio digitali e l'accesso ai servizi informatici da parte dei cittadini. La semplificazione riguarda anche la conservazione di informazioni e documenti in formato digitale, nel rispetto delle norme di tutela della *privacy*. Il recente passato e le difficoltà create dall'emergenza coronavirus, non ancora conclusa, impongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di sviluppare sistemi idonei a garantire ai dipendenti l'esercizio del lavoro a casa in sicurezza ed efficienza. A tal fine, il Governo vuole instaurare misure di semplificazione e coordinamento dell'attività potenziando il Dipartimento della trasformazione digitale. Il passo successivo al potenziamento dello *smart working* sarà l'introduzione di un codice di condotta tecnologica, con regole omogenee valide per tutte le ramificazioni della pubblica amministrazione. Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte dell'amministrazione di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale. L'articolo 33 sanziona i dirigenti responsabili di inadempimento e prevede l'obbligo, per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti. Con il Titolo II, interveniamo sulla semplificazione del provvedimento amministrativo. Infatti, l'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, la legge n. 241 del 1990, in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa. Viene inoltre previsto l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché di aggiornare i termini di quelli di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata. Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la piena operatività dei meccanismi di silenzio-assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine. Un secondo gruppo di disposizioni introduce misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo. Centrali, in questo decreto, sono anche la tutela dell'ambiente e i progetti inerenti all'energia rinnovabile. Il Titolo IV, infatti, contiene disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, ambiente e *green economy*. L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno degli investimenti, la cosiddetta Nuova Sabatini. In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogato in un'unica soluzione; inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, dell'economia e delle finanze, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma d'investimento, nonché la possibilità di utilizzo di fondi europei. L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al codice unico di progetto, in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano e attuano progetti d'investimento; dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. Stabilisce infine che i sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione. L'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo. Prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale, il SIAN, sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche geospaziali. Apporta modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche quelle alimentari e mangimistiche. Interviene in materia di sanzioni in caso di sospensione ed esclusione dal metodo di produzione biologica e introduce la comunicazione individuale - al posto dell'attuale, espletata attraverso la pubblicazione sul sito dell'INPS - degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. L'articolo 47, infine, reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso un'accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ed atti alle attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per l'attenzione.

C'è un motivo sostanziale per cui sarebbe opportuno che l'Assemblea, in via pregiudiziale, non procedesse con l'esame e l'approvazione di tale normativa, cioè il fatto che un decreto-legge così corposo, che dovrebbe dare una svolta reale, vera e concreta alla burocrazia del nostro Paese lo sappiamo benissimo - ci costa 57 miliardi di euro, pari, tanto per capirsi, alla metà del debito che abbiamo fatto con gli ultimi scostamenti

C'è anche un'altra questione che dovrebbe far riflettere. Questo è un decreto-legge semplificazioni a costo zero e, conseguentemente, non costituisce un'opportunità politica

Questo è il terzo elemento che, a mio avviso, dovrebbe indurre a valutare attentamente l'opportunità politica di non andare avanti in via pregiudiziale con l'esame di questo testo. capisco che c'è molta stanchezza, perché davvero il Senato ha lavorato sempre, e con ritmi incredibili, durante tutta l'estate, però cerchiamo di avere un altro po' di pazienza e ascoltare la senatrice Modena.

come se fosse tutto sparpagliato nella sabbia, da imporre una riflessione seria e

pregiudiziale con riferimento all'articolo 93 del Regolamento del Senato.

Di fronte alla scelta che è stata fatta attraverso le varie opzioni del decreto-legge semplificazioni (gli interventi sugli appalti pubblici per gli acquisti la velocizzazione delle procedure nella pubblica amministrazione, rispetto agli appelli che ci sono giunti trasversalmente da tutti i rappresentanti sociali del nostro Paese), non nascondiamo lo stupore lo stupore per una questione pregiudiziale che, se dovesse passare, determinerebbe un rallentamento di tutto quello che finora non solo abbiamo detto in ogni sede, ma ci è stato chiesto, ovvero la velocizzazione e la sburocratizzazione

tutti gli interventi economici a sostegno delle iniziative imprenditoriali in difficoltà a causa del Covid. Poi, visto che stiamo esaminando una questione pregiudiziale, non si capisce come una previsione possa superare le ragioni di costituzionalità,

peraltro, si scrive anche che i provvedimenti, che non sarebbero d'immediata attuazione, creerebbero un impatto negativo sugli obiettivi.

fino a dicembre 2021 tutte le procedure, in particolare per gli investimenti pubblici. Quindi non si capisce quali siano questo rallentamento e questo impatto immediato sulle iniziative economiche del nostro Paese. Nel quadro delle difficoltà che stiamo descrivendo è però certamente esilarante

Facciamo fatica a immaginare come questo possa avvenire: eventualmente è il codice degli appalti derogato che potrebbe creare contenziosi, non la deroga delle procedure.

una pregiudiziale per bloccare tutto. In realtà, il decreto semplificazioni interviene sulle procedure in essere con strumenti, soluzioni e categorie già sperimentati e noti agli operatori economici, quindi non vi è contraddittorietà rispetto alle previsioni

per le attività imprenditoriali del nostro Paese, ragione per la quale diciamo che l'urgenza è nelle cose. Se passasse invece questa pregiudiziale, tutto tornerebbe in bilico, come prima: non velocizzeremmo nulla e non daremmo alcuna risposta alle richieste pervenute da tutte le parti, che ci sono state confermate nelle tantissime audizioni svolte sul provvedimento,

la seguente comunicazione: *Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2,

senatori, ringrazio tutti voi per questa ulteriore occasione di confronto in un passaggio che ritengo particolarmente delicato dell'evoluzione epidemiologica nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. Considero, com'è noto, ogni passaggio parlamentare mai rituale o formale ma occasione utile per raccogliere spunti e suggerimenti dentro una dialettica che mi auguro possa essere sempre la più proficua possibile, nella consapevolezza che la discussione, anche se aspra, rende sempre più forte la nostra democrazia. Rispetto al mio ultimo passaggio in quest'Aula che - voglio ricordarlo - è avvenuto il 10 agosto, il quadro epidemiologico europeo si è giorno dopo giorno significativamente deteriorato e anche nel nostro Paese, in Italia, pur se in un quadro lontano da quello dei Paesi europei che incontrano maggiori difficoltà, abbiamo riscontrato una graduale salita del numero dei contagi. Voglio iniziare la mia comunicazione con i dati, perché come sempre i dati, i numeri, ci illustrano lo scenario in maniera molto più semplice e lineare:

23, un dato molto simile a quello della Germania che, ad oggi, è tra i migliori nel contesto europeo. Nel frattempo, a livello mondiale, la situazione si è ulteriormente complicata. Siamo ormai arrivati a 25.700.000 casi con 857.000 decessi. Questi numeri ci dicono alcune cose che dobbiamo provare a leggere e ad analizzare tutti insieme. *In primis* ci dicono che il *lockdown* nel nostro Paese ha funzionato e che il comportamento degli italiani e le misure del Governo nazionale, come quelle dei governi regionali, sono riuscite a piegare la curva e ci consegnano ancora un significativo vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei. Io penso che questo sia un risultato importante che dobbiamo saper riconoscere insieme. È un risultato di tutti, che ci viene attribuito anche sul piano internazionale. Non è un risultato del Governo, non è il risultato delle Regioni. A me piace dire sempre che è un risultato di tutte le nostre istituzioni repubblicane, è un risultato della nostra comunità nazionale conseguito in una prova durissima, chiaramente non ancora vinta,

alla resilienza del nostro Servizio sanitario nazionale e, in modo particolare, alle donne e agli uomini che vi operano a cui va e andrà sempre la nostra più sentita gratitudine. I numeri che sono cresciuti anche nel nostro Paese nelle ultime settimane, negli ultimi venti giorni, hanno risentito sicuramente anche di una crescita dei test e del numero dei tamponi che sono stati effettuati. Voglio ricordare che durante l'ultima settimana abbiamo sfiorato il dato di 100.000 tamponi in un solo giorno, giorno, anche alla luce di una significativa intensificazione del lavoro negli aeroporti dove, rispetto agli arrivi dai Paesi a rischio (su questo tornerò in seguito), si stanno iniziando ad usare anche i test rapidi antigenici. C'è una novità rispetto alla drammatica stagione che abbiamo vissuto nei mesi di marzo e di aprile. Il nostro sistema di monitoraggio, quello costruito settimanalmente con l'Istituto superiore di sanità e con le Regioni, ha segnalato negli ultimi sette giorni una media di età dei contagiati di ventinove anni. Penso che questo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo naturalmente riflettere, anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo.

estive, della questione dei giovani del nostro Paese e dell'innovazione che comporta rispetto ai mesi precedenti. Più volte, anche pubblicamente, chiesto una mano ai nostri ragazzi: lungi da noi ogni forma di demonizzazione, che non avrebbe alcun senso, ma è vero che dobbiamo chiedere, soprattutto ai nostri giovani, di darci una mano. È senz'altro vero che il virus tra le generazioni più giovani fa meno male rispetto all'impatto che esso ha naturalmente sulle generazioni più avanti negli anni, ma è altrettanto vero giovani continuano a essere comunque uno strumento di diffusione del virus, e questo può essere pericoloso, qualora il virus dovesse estendersi in modo particolare ai genitori e ai nonni, che pagherebbero un prezzo molto più alto. Alla luce di questo quadro, ai giovani, ma più in generale a tutti i nostri concittadini, continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali che sono rimaste,

Le tre regole si sostanziano nell'uso corretto delle mascherine, nel distanziamento di almeno un metro e nel rispetto delle norme igieniche fondamentali, a partire dal lavaggio delle mani. Sono tre pilastri veri e propri su cui tutta la comunità scientifica internazionale è profondamente d'accordo: non c'è nessun Paese del mondo in cui la comunità scientifica dissenta rispetto alla necessità di osservare queste tre regole fondamentali. opinione, quindi, è che su questo non dobbiamo assolutamente dividerci: non è materia di contesa politica, non c'entrano la destra, la sinistra o altro. Sono tre regole essenziali che ci devono accompagnare in questa fase importante di convivenza con il virus. Dal 6 agosto, l'ultimo giorno in cui sono stato in quest'Aula per un'informativa, ho firmato due ordinanze che ritengo essere state importanti, anche se, com'è noto, ogni ordinanza comporta sempre in qualche modo un sacrificio, un prezzo che la nostra comunità decide di pagare. La prima ha riguardato l'estensione di test obbligatori a persone che negli ultimi quattordici giorni sono stati in Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Questi test possono essere effettuati o prima della partenza dal Paese di provenienza oppure nei luoghi di arrivo - penso ai porti, agli aeroporti e il nostro sistema si è organizzato in maniera rapida e significativa per predisporre questi presidi nei luoghi di arrivo - o, ancora, nelle quarantotto ore successive presso le nostre aziende sanitarie. Credo che queste misure siano state importanti e in questo passaggio in Aula qui in Senato - sarò più tardi alla Camera - voglio rendere nota una proposta che come Governo italiano stiamo portando all'attenzione di tutti gli altri Paesi europei. La proposta parte da un'idea molto semplice: quando assumiamo una misura di maggiore controllo dei nostri confini e degli arrivi nel nostro Paese non compiamo mai un atto ostile nei confronti di quel Paese, è un atto che vuole semplicemente aumentare il livello di sicurezza. La nostra proposta come Governo italiano agli altri Paesi europei, che porterò in modo particolare il 4 settembre alla riunione dei Ministri della salute dell'Unione europea, è che si possa costruire un meccanismo di reciprocità tra i Paesi. Proprio per eliminare dal tavolo questo elemento di ostilità che in alcuni casi viene così interpretato nelle relazioni tra i Paesi, credo che la cosa più intelligente sia condividere un meccanismo di reciprocità. Dobbiamo convivere con questo virus ancora per un tempo significativo. Stiamo investendo sul vaccino (lo dirò alla fine) e sulle cure con tutte le energie che abbiamo, ma è chiaro che di fronte a noi abbiamo nella migliore delle ipotesi ancora alcuni mesi di convivenza. Se proprio non vogliamo stringere le relazioni tra i Paesi, se non vogliamo correre il rischio di arrivare ad ulteriori momenti di riduzione della mobilità tra i Paesi, l'idea di fare test nei principali aeroporti del nostro Continente ci sembra un'idea giusta, che in uno spirito collaborativo e inclusivo ci può portare - crediamo - ad ottenere risultati giusti. La seconda ordinanza che ho firmato durante queste settimane, in modo particolare il 16 agosto, riguarda la sospensione delle attività di ballo, non solo nelle discoteche ma anche in luoghi affini, e l'utilizzo obbligatorio delle mascherine all'aperto dopo le ore 18 nei luoghi dove c'è rischio di assembramento. Voglio utilizzare questo passaggio in Parlamento per chiarire che il Governo nazionale nei suoi provvedimenti formali non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche, ma com'è noto dal 16 maggio le Regioni hanno avuto la facoltà non solo di applicare misure più restrittive (facoltà che era già prevista nella fase precedente e più drammatica dell'emergenza), ma anche di mettere in campo misure meno restrittive. Dentro quest'ambito alcune Regioni hanno utilizzato queste facoltà. Permettetemi ancora una volta di ribadire che ogni ordinanza comporta evidentemente un sacrificio e un costo per il nostro Paese, ma ritengo che queste ordinanze siano state giuste e opportune e che ci consentono di conservare quel vantaggio rispetto ad altri Paesi di cui ho provato velocemente a parlare. e il suo obiettivo fondamentale è in questo momento quello della riapertura delle scuole e anche tutti i sacrifici che stiamo tenendo ancora in piedi hanno quello come obiettivo fondamentale. Penso che chiudere le scuole abbia rappresentato per tutti noi, per me in modo particolare, la scelta più difficile e voglio dire che oggi riaprirle è davvero la nostra priorità assoluta su cui stiamo impegnando tutte le energie di cui disponiamo. Permettetemi in questa sede di ricordare che stiamo parlando di un grande tema di carattere mondiale: sono stati 190 i Paesi del mondo che durante questi mesi hanno sospeso le attività scolastiche. In questi 190 Paesi gli studenti coinvolti sono stati 1,6 miliardi: stiamo quindi parlando di numeri che - come vedete - hanno una portata di natura planetaria. Mi piace ricordare solo in un istante

copresiedere, che ha avuto come obiettivo fondamentale proprio quello di provare a condividere alcune regole essenziali per la riapertura delle scuole. All'esito di questa riunione

area abbiamo deciso di costruire una piattaforma permanente per mettere a sistema le migliori esperienze e le nostre conoscenze e anche per poter aggiornare le linee guida che stiamo costruendo sulla base di relazioni innovative che possono arrivarci dal mondo scientifico e dalle nuove conoscenze. Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e lo faranno in sicurezza. Già ieri è stato molto bello poter vedere le immagini di una parte dei giovani del nostro Paese che, per i corsi di recupero, hanno ricominciato ad entrare negli istituti scolastici. Voglio ricordare in questa sede che pochi giorni fa abbiamo approvato, in Conferenza unificata, con l'opinione unanimemente favorevole delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani, il documento dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute sulle linee guida per la gestione dei casi Covid-19 e dei focolai Covid-19; si tratta di un documento che ci consentirà, senza alcuna differenziazione di natura territoriale, di gestire gli eventuali casi e gli eventuali focolai. Io penso che avere su questo un elemento di piena omogeneità nel nostro Paese sia sicuramente un fatto positivo e importante. Sulla base delle linee guida, che - ripeto - abbiamo approvato all'unanimità con tutte le Regioni, i Comuni e le Province del nostro Paese, sta partendo proprio in queste ore un corso di formazione, organizzato dall'Istituto superiore di sanità, rivolto alla nostra popolazione studentesca e, in modo particolare, al personale che lavora nelle scuole, ma anche al personale medico, per poter essere pienamente allineati rispetto agli obiettivi che stiamo costruendo. Come ho avuto già modo di dire in questa Assemblea in altri passaggi, a mio avviso la chiave fondamentale rispetto alla riapertura delle scuole consiste nel ricostruire una relazione organica tra scuola e Servizio sanitario nazionale. Questa relazione è esistita in una fase della storia del nostro Paese: nel 1961 il Parlamento italiano approvò una norma che riguardava la cosiddetta medicina scolastica. Questa rete di relazioni, questo momento di contatto costante tra scuola e servizio sanitario nazionale si è poi andato, un po' alla volta, perdendo; in modo particolare, negli anni Novanta se ne è persa traccia. Ebbene, credo che dobbiamo puntare su questo: ricostruire una relazione organica e strutturata, costante e permanente, tra il servizio sanitario nazionale e il sistema scolastico del nostro Paese. Se ci saranno - come sarà abbastanza naturale - dei casi positivi nelle scuole, saranno i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie territoriali

di positività. Il messaggio di fondo che vorrei trasmettervi è che, rispetto a casi di positività, non lasceremo soli i nostri presidi e i nostri insegnanti, ma ci sarà una presenza significativa dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, perché è giusto che chi ha la competenza, la storia, le esperienze e ha già operato costantemente rispetto alla necessità di affrontare questo virus possa mettere queste competenze a disposizione delle scuole. Lo stesso lavoro che si sta facendo in queste ore con i test sierologici sugli insegnanti e su tutto il personale scolastico ha esattamente questo significato: rafforzare la relazione tra mondo della scuola e mondo della sanità. Permettetemi di esprimere gratitudine a tutti i medici di medicina generale che stanno dando una mano nell'ambito di questo lavoro *(Applausi)*, che è abbastanza unico

assolutamente importante. Nelle ultime ore il Comitato tecnico-scientifico ha anche discusso di un tema di particolare importanza, che ha toccato una preoccupazione diffusa tra le famiglie, e cioè la necessità di un corretto utilizzo delle mascherine. Come ho già detto, le mascherine sono uno strumento fondamentale che dovremo tenere in questa fase di convivenza. Il Comitato tecnico-scientifico nelle ultime ore ha definito le sue raccomandazioni sull'utilizzo corretto delle mascherine a scuola. Provo a dirla così: le mascherine a scuola sono obbligatorie; proprio perché sono fondamentali, a scuola si va con la mascherina, ma poi distinguiamo due momenti: quelli dinamici, in cui ci sono rischi concreti per i nostri studenti di poter avere contatti più ristretti, a meno di un metro di distanza con altri studenti,

Nel momento statico la mascherina, che è obbligatoria negli altri momenti, può essere abbassata. Questa misura può essere rivista nel caso di situazioni epidemiologiche particolarmente delicate, ma saranno solo le autorità sanitarie a disporle e a valutarle in modo corretto. Permettetemi di dire - penso sia un fatto importante - che siamo l'unico Paese in Europa, e credo anche nel mondo, che metterà a disposizione come istituzioni pubbliche 11 milioni di mascherine *(Applausi)* per ciascuno dei nostri studenti e per tutto il personale scolastico. Saranno mascherine chirurgiche distribuite gratuitamente e di questo voglio ringraziare il prezioso lavoro del nostro commissario straordinario Arcuri. Ancora, il 31 agosto, come è noto, la Conferenza unificata, sempre con un parere all'unanimità delle Regioni, delle Province e dei Comuni del nostro Paese, ha approvato le nuove linee guida sul trasporto pubblico locale. Anche in questo caso abbiamo provato a conciliare due necessità che dobbiamo tenere insieme, e non è mai facile - lo dico con grande sincerità - trovare un equilibrio tra queste necessità: avere una cautela sanitaria rispetto a un virus che ancora c'è e con cui dobbiamo fare i conti, ma anche la necessità, che emergeva in modo particolare dai nostri Comuni, dalle nostre Province e dalle nostre Regioni, di provare a garantire un trasporto pubblico per tutti. Credo che sia stato fatto un lavoro importante e che queste linee guida possano consentirci di raggiungere un equilibrio positivo. Ancora sulle scuole, permettetemi di ricordare che in queste settimane è stato definito un investimento diretto senza precedenti anche in termini di risorse economiche, umane e strumentali. I problemi della scuola non sono pochi e, come è noto, non vengono da vicino, ma da lontano: ad esempio, la questione dell'affollamento delle classi non nasce con il Covid. Ci sono problemi e temi che riguardano la scuola che vengono da stagioni precedenti, però non possiamo nasconderci quello che in queste ore si sta facendo: 2,9 miliardi di euro messi a disposizione della ripartenza delle nostre scuole; 97.000 immissioni in ruolo che sono in corso, quindi un numero significativo di nuovi insegnanti e di nuovo personale che mettiamo a disposizione dei nostri studenti e delle nostre famiglie; 2,4 milioni di nuovi banchi. Voglio provare in questa sede a dare un messaggio molto chiaro e molto netto: la riapertura delle scuole è una grande priorità; credo che sia la più grande priorità oggi per il nostro Paese. Non è una priorità del Governo, delle Regioni o dei Comuni e delle Province, che pure stanno lavorando con noi ogni giorno gomito a gomito. Credo che la riapertura delle scuole sia la più grande priorità per tutta la nostra comunità nazionale. E allora dico: lavoriamo insieme per recuperare lo spirito che ci ha accompagnato nei mesi più difficili, ossia nei mesi di marzo e di aprile, quando il Paese si è unito. Penso che dobbiamo recuperare esattamente quello spirito e che serva un nuovo patto che coinvolga tutti, nessuno escluso: Governo, Regioni, Parlamento, ma anche e soprattutto studenti, presidi, genitori, personale sanitario. È una sfida che si vince solo uniti; non servono inutili divisioni o inutili strumentalizzazioni. Ancora, consentitemi, in chiusura, un veloce aggiornamento su quella che ritengo essere una partita decisiva per provare a chiudere definitivamente questa sfida della gestione del Coronavirus e cioè la vicenda che riguarda i vaccini. che sul vaccino tradizionale, quello antinfluenzale, abbiamo la necessità di costruire quest'anno una campagna più forte rispetto a quella fatta negli altri anni, proprio perché i sintomi sono simili e questo potrebbe provocare difficoltà al nostro Servizio sanitario nazionale. le Regioni hanno fortemente irrobustito la loro offerta del vaccino antinfluenzale e ieri si è tenuta una riunione, aprendo un tavolo con i farmacisti italiani, esattamente su questa materia. Per quanto riguarda invece il vaccino anti-Covid, voglio ricordare come l'Italia sia davvero in prima linea in questa battaglia. L'alleanza che abbiamo costruito già nel mese di giugno con Francia, Germania e Olanda ha consentito di spingere la Commissione europea ad una forte accelerazione delle politiche rispetto alla potenzialità di avere un vaccino sicuro nel più breve tempo possibile. Com'è noto, nelle ultime ore è stato reso definitivo in maniera ultimativa il contratto tra la Commissione europea ed AstraZeneca e quel contratto parte esattamente dall'intesa fatta da Italia, Germania, Francia e Olanda con questa importante azienda. Stiamo parlando, chiaramente, di un candidato vaccino, quindi c'è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto c'è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come un vaccino sicuro e in grado di raggiungere l'obiettivo per cui è stato ricostruito, saranno già disponibili entro la fine del 2020, quindi è giusto continuare ad investire su questo, con tutte le energie che abbiamo. Mi piace ricordare che in questo vaccino di AstraZeneca c'è un pezzo d'Italia che è pienamente protagonista, perché il vettore virale viene prodotto presso l'IRBM di Pomezia e perché l'infialamento di questo vaccino avverrà presso la Catalent di Anagni. quindi, come vedete, è pienamente protagonista e credo che questo sia un fatto di particolare rilievo per il nostro Paese. Permettetemi ancora di ricordare che alla fine del mese di agosto, negli ultimi giorni, è anche stata avviata la sperimentazione sull'uomo del vaccino di ReiThera, che è un vaccino tutto italiano e anche da questo punto di vista credo che ci siano elementi per esprimere profonda gratitudine ai nostri scienziati, ai nostri ricercatori che non stanno facendo mancare il loro contributo a questa importante sfida mondiale.

per qualche giorno, ma sono ottimista che nel prossimo decreto ci possa essere una soluzione riguardo, ad esempio, alla richiesta di ricongiungimento delle coppie binazionali. Su questo avevo risposto in Aula ad una interrogazione della senatrice Unterberger

tutti i verbali del Comitato tecnico-scientifico. La linea del Governo è stata sin dall'inizio una linea di massima trasparenza, stiamo lavorando perché questi verbali, nei quali non c'è assolutamente nulla che non possa essere reso noto all'opinione pubblica, possano essere pubblicati. Infine, permettetemi di dire che ascolterò con grandissima attenzione, come ho sempre fatto, l'indirizzo del Parlamento e sono sicuro che anche in questo passaggio autunnale che sta per arrivare l'Italia saprà essere all'altezza della sfida che abbiamo di fronte a noi.

però di tutta evidenza che a queste comunicazioni manca del tutto un approccio stringente, atto a governare le priorità in materia sanitaria che avrebbero già dovuto essere affrontate da mesi, quali misure fondamentali da adottare durante lo stato di emergenza pandemica in punto di profilassi internazionale, prevenzione e contenimento della circolazione del virus*,* quale precondizione di sistema nazionale non ulteriormente rimandabile. Non mi soffermerò su quanto ha detto relativamente alla scuola e ai trasporti, perché sono sicuramente fuori moda, ma ritengo doveroso parlare solo di quello che so. È palese che arrivare impreparati al periodo autunnale, con un'eventuale seconda ondata, anche importata da altri Paesi, non sarebbe ammissibile. che il Governo voglia tenere fede alla dichiarazione del presidente Conte, che ha affermato che non ci sarà mai più una chiusura totale.

ci saremmo aspettati che, ad esempio, fosse fatto obbligo a tutti gli erogatori accreditati a contratto che, prima di somministrare

Questo sarebbe dovuto essere uno dei pochi argomenti che potevano giustificare il proseguo dello stato di emergenza sanitaria, incidendo su libertà fondamentali per il bene superiore della tutela della salute della collettività, nell'obiettivo della migliore salvaguardia della salute dei singoli mediante azioni mirate di prevenzione e regimi di protezione differenziati e crescenti per età e fragilità,

dove il rischio maggiore riguarda anziani e malati cronici con almeno una patologia preesistente. Fornendo quindi come Protezione civile, a tutti gli erogatori della rete i *test* diagnostici approvati e validati nel quadro di un programma straordinario stringente di attività di sorveglianza e di *screening* delle popolazioni ad alto rischio attraverso la combinazione di sierologia e tamponi virologici. Queste sarebbero state le comunicazioni che ci saremmo attesi, non generiche dichiarazioni di principio. Non il perpetuarsi di un meccanismo di trasferimento delle responsabilità e relative risorse economiche indifferenziate sul livello territoriale, senza tracciabilità degli impieghi, rimettendo tutto alla buona volontà di chi è a vicariare competenze altrimenti dello Stato.

che avrebbero limitato di molto le incongruenze, e non solo nel settore sanitario e scolastico, che sono i settori a maggiore vulnerabilità, perché non volevamo e non vogliamo credere che questo Governo, nonostante tutto, voglia intenzionalmente arrecare nocumento al sistema Paese, ma non ne abbiamo trovato traccia né nel decreto-legge semplificazioni né nel decreto-legge agosto. Né tantomeno nelle sue comunicazioni, posto che ci saremmo aspettati che ci avesse illustrato il tanto atteso piano nazionale emergenziale integrato di misure di controllo, di prevenzione e preparazione anti pandemia. di monitoraggio continuo che investa in ricerca epidemiologica e clinica, concentrando gli sforzi di investimento e di adattamento al sistema anche sul versante dell'innovazione per il riconoscimento tempestivo e l'interruzione precoce delle catene di contagio quale risposta più efficace per la protezione della popolazione.

acquistando e mettendo a disposizione quanto serve e quando serve secondo l'effettiva incidenza del rischio. Spendere senza precisi programmi validati vuol dire sovvertire, anche in sanità, il già indigesto principio della sinistra "tassa e spendi" in prima spendi e poi tassa. che questa involuzione non sfuggirà nella sua gravità agli italiani quando saranno chiamati alle urne.

Ministro, si consuma per l'ennesima volta questa sorta di interposizione fittizia di Speranza, che non è solo un auspicio di speranza che naturalmente condividiamo, ma è proprio il fatto che ci viene frapposto il suo *speaking* - mi consenta, Ministro - un po' democristiano, che tradisce in parte le sue origini

Capisco la necessità di coprire tutto ciò che non va - poi magari ce lo diremo nel prosieguo dell'intervento e degli interventi

a tanti suoi colleghi di Governo o anche ai segretari dei partiti che lo sostengono, a cominciare da Zingaretti, che dice invece che il Governo ha salvato l'Italia rispetto a non si capisce bene cosa, visto che il virus l'abbiamo preso, l'abbiamo digerito, l'abbiamo gestito, lo abbiamo sopportato e, probabilmente, in qualche misura, avendolo preso per primi, ne stiamo faticosamente uscendo altrettanto per primi. Va però ricordato che ciò è stato grazie all'impegno costante, continuo ed eroico di una categoria sociale, quella degli operatori del Servizio sanitario nazionale, e alla misure di banale distanziamento, come lavarsi le mani, proteggersi la bocca, restare a casa, lasci dire - non serve contenere in un'azione di Governo, ma basta riepilogare in provvedimenti di buon senso. vorremmo affrontare nel merito un periodo, che ci ha visto per oltre sei mesi impegnati fortemente a a contrastare un'epidemia, che è entrata nel nostro Paese con fin troppa facilità. Come ricordiamo nel nostro atto di indirizzo, in tempi utili e non sospetti, senza avere a disposizione i verbali che invece aveva a disposizione il Governo, come oggi e nei giorni scorsi è stato riepilogato dagli organi di stampa, e che prefiguravano addirittura casi di mortalità

auspicavamo, già nei mesi di marzo e di febbraio, misure contenitive atte a proteggere i confini, a testare la presenza del virus nei viaggiatori provenienti dalle zone a rischio e ad adottare fin dall'inizio, come ricordiamo nella nostra proposta di risoluzione, misure di contenimento, come le mascherine e il distanziamento e di igiene, come lavarsi le mani.

con un attimo di senso di responsabilità in più, riconoscendo che alcuni errori sono stati compiuti, che i protocolli iniziali di terapia e cura erano completamente sballati, che alcuni percorsi - mi riferisco al plasma iperimmune e all'idrossiclorochina - non si capisce bene a quale titolo e perché ancora ad oggi sono contrastati e sono stati utilizzati con ritardo e non a sufficienza. In sostanza, oggi dovremmo affrontare tutti questi temi fuori dalla dialettica buonista

mi perdoni, signor Ministro - nei fatti non esiste, perché il contributo delle istituzioni parlamentari è pari a zero, perché tutti i provvedimenti vengono approvati con l'apposizione della questione di fiducia, perché lo spazio riservato all'azione emendativa e migliorativa dei provvedimenti è pari a zero, perché poi le cose proposte magari vengono affrontate nei provvedimenti successivi, camuffandole in altro modo, pur di non dare accesso (non dico ragione, ma almeno accesso) alle proposte di più banale buon senso. Quindi, rispetto a tutto questo, un po' di preoccupazione io la manifesto, anche a dispetto del suo incedere rassicurante.

molto radicalmente, a cominciare evidentemente dall'età media dei contagiati, ma non solo. Penso anche alle catene di trasmissibilità, che

quali e quanti di questi sono in grado di trasmettere? Lo sappiamo? Esiste uno studio, un'analisi, un'indagine, un'asticella messa a un livello che misuri la carica virale

i non sintomatici vanno trattati a partire dalla loro capacità di trasmettere il virus. Se uno è non sintomatico, cioè sta bene, e non è capace di trasmettere, allora anche le misure di contenimento vanno tarate in questo senso, perché è difficile costringere queste persone a stare a casa. C'è gente che è positiva per due, tre o quattro tamponi e non ha niente;

Che succede? Lo possiamo sapere? Ce lo dirà in qualche modo la comunità scientifica, attraverso questo famigerato e fantomatico Comitato tecnico-scientifico, del quale aspettiamo di leggere i copiosi verbali, ivi compresi gli allegati? colleghi, ci suggerisce alcune indicazioni. Non che siamo così ottimisti sul fatto che prendiate per buone tali indicazioni, ci mancherebbe; però comunque è dovere nostro rappresentarle, se non altro a beneficio è che noi ancora oggi, a sei mesi abbondanti, continuiamo a tracciare i sintomi. Noi ancora oggi andiamo dietro ai sintomi, sapendo che sei o sette su dieci sono senza sintomi. Noi oggi ancora partiamo dal sintomo. Dobbiamo approfondire l'indagine per individuare i non sintomatici, sì o no?

reso disponibile copiosamente, coinvolgendo le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale e tutte le strutture di prevenzione. Tutti sono pronti a fare questo approfondimento di indagine e questo è quanto dobbiamo fare. Seconda cosa:

Voi avete usato uno strumento universalmente considerato illegittimo in una fase di grave emergenza; va bene, l'avete fatto e ve ne siete presi la responsabilità. Non lo dico io, lo dicono i costituzionalisti; c'è una lunga serie di costituzionalisti che lo dicono, anche gente che non è certamente di Fratelli d'Italia, né del centrodestra. Però questo è stato fatto in una fase emergenziale, che nessuno nega essere stata emergenziale. Oggi quell'emergenza non c'è.

percorsi normali; ripristiniamo la gerarchia delle fonti. E poi basta con la proroga dell'emergenza. Non c'è emergenza o, perlomeno, non c'è un'emergenza tale da giustificare gli stessi strumenti.

Noi oggi abbiamo cominciato ad analizzare il decreto agosto, i cui effetti si esauriranno a fine anno. Non è possibile continuare a mettere in campo provvedimenti che hanno un respiro di due o tre mesi: la sanità ha bisogno di provvedimenti di sistema anche alla luce dell'emergenza che c'è stata.

poiché sono cittadini molto giovani e - mi auguro - in buona salute, non sono come i nostri cittadini che purtroppo non ci sono più e che presentavano una comorbilità che ha portato al decesso di troppe persone per questa emergenza.

c'è un paradigma che sposta sul territorio una prevenzione che è importante. Devo dire che il Covid ha accelerato tutte le titubanze e le ritrosie accumulate negli anni e nel tempo

e stiamo mettendo in pratica cose che prima si pensava non avessero la stessa efficacia. Abbiamo trovato invece efficacia anche in questi sistemi e non meno nei sistemi innovativi della telemedicina. telemedicina. Anche questo è un paradigma cambiato: pensiamo al telemonitoraggio, alla televisita, alle ricette elettroniche e addirittura all'utilizzo dei sistemi di applicazione dei nostri cellulari. Quindi, come vedete, ci

quindi tutto quello che si sta facendo. Va anche bene il fatto che lei, signor Ministro, abbia preso in mano una situazione che si stava aggravando ulteriormente, tenendo in considerazione che le Regioni hanno un

comparazione con gli altri Paesi per quanto riguarda le linee guida per la scuola. Prioritariamente e giustamente io sono d'accordo sul fatto che debba riaprire, avendo però un'interlocuzione a livello europeo per lo meno per sapere che cosa fanno gli altri Paesi. Noi ci siamo mossi in una certa maniera per tutelare e garantire la sicurezza delle nostre famiglie. anche gli altri Paesi, ma abbiamo visto quanti di essi sono dovuti ritornare sui loro passi. Quindi noi, in tutta sicurezza, dobbiamo garantire, soprattutto in ambito scolastico, certezza e garanzia che i protocolli vengano applicati

padri e madri, che si sentissero isolati e soli. Questo per me è molto importante. Per tutto il resto, signor Ministro, credo che stiamo andando dalla parte giusta. Controlliamo, ovviamente, e monitoriamo quello che si sta facendo da adesso in poi. La sfida dell'apertura della scuola è importantissima e io credo

Non mi riferisco neanche soltanto a quella presentata ai primi di maggio circa le circolari emesse dal suo Ministero che bloccavano da più di un mese le autopsie ai pazienti deceduti per Covid, cosa che sembrava molto strana visto che solo grazie alle autopsie è stato possibile capire il meccanismo di questa terribile malattia. Fortunatamente, poi, nel mese di giugno sono state sbloccate. Avevamo presentato anche un'interrogazione sui test sierologici. Conosciamo tutti il *flop* dei testi sierologici perché su 190.000 persone che si pensava di coinvolgere in due settimane,

Ministero e ulteriori fondi elargiti dalle donazioni volontarie. Sapevamo perché sarebbe stato un *flop*: non era possibile far trascorrere troppi giorni tra un test sierologico apparentemente positivo e il tampone, quindi le persone non hanno aderito. Anzi, vorrei sollecitare anche la risposta ad un'interrogazione che Forza Italia ha depositato oggi affinché possano essere eseguiti i test sierologici su tutti gli scrutatori e tutti i presidenti delle sezioni elettorali. Non ho mai avuto risposta a una mia interrogazione sui lavoratori fragili, e infatti il Governo se n'è dimenticato, perché nelle disposizioni che prorogavano lo stato di emergenza fino al 15 ottobre manca sorprendentemente la norma che consentiva ai lavoratori con una disabilità grave, malati di tumore, trapiantati, affetti da malattie rare e quindi immunodepressi, di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro equiparato al ricovero ospedaliero. Sono state date mance e mancette a destra e a sinistra, ma sui lavoratori fragili c'è stata una disattenzione imperdonabile. Ci auguriamo, Ministro, che lei possa risolvere al più presto questa incresciosa situazione. Nessuna risposta, inoltre, è stata data ad una mia interrogazione presentata mesi fa sulla mancanza di un piano pandemico nazionale per poter contenere le possibili situazioni emergenziali, anche sugli sbarchi degli immigrati. L'ultimo piano pandemico risale al 2010 e poi più niente. Ora, gli italiani usciti da qualche mese dal *lockdown* e ancora alle prese con restrizioni prudenziali sia imposte dalla pandemia e dalle disposizioni, ma anche dalla responsabilità

Il ministro Azzolina ha fatto ricadere tutte le responsabilità sui presidi per gestire il buon andamento della didattica degli istituti. Credo che tutti si aspettino poche parole che non si smentiscano un giorno dopo l'altro e linee guida chiare. Detto questo, sappiamo quante situazioni urgenti il nostro Paese e il nostro sistema sanitario hanno dovuto affrontare. Molti ospedali italiani, travolti per mesi dall'ondata di ricoveri, hanno interrotto le prestazioni erogate per i pazienti affetti da altre gravi patologie. Sono stati interrotti gli *screening* oncologici, essenziali per individuare precocemente i tumori e intervenire tempestivamente; secondo un sondaggio promosso da un'associazione, più del 36 per cento di pazienti ha lamentato la sospensione di esami e visite di *follow-up*. rinviati per mesi anche gli interventi chirurgici; dai dati registrati in 54 strutture cardiologiche universitarie i ricoveri per infarto si sarebbero dimezzati, ma la mortalità per infarto è triplicata. Questi sono i dati anche della Società italiana di cardiologia. Non più confortanti certo sono i dati relativi alla cura delle malattie rare: secondo l'Istituto superiore di sanità oltre il 50 per cento dei pazienti ha dovuto interrompere il proprio percorso terapeutico.

Io sono consapevole che le misure di prevenzione impongono il distanziamento tra i pazienti, separatori fisici e igienizzazione, ma il timore è che non si adottino con tempestività misure opportune per programmare l'attività ospedaliera rispondere in modo adeguato ai tanti italiani che da mesi aspettano prestazioni sanitarie essenziali o addirittura salvavita. È inutile che continui con questo triste elenco. Sappiamo come le liste d'attesa siano drammatiche (lo erano già prima e lo sono ancora di più adesso). Abbiamo visto nel decreto agosto che sono state prese delle misure e speriamo che possano essere efficaci, efficaci, perché le persone non possono più aspettare. Credo sia necessario intervenire proprio per evitare ricadute catastrofiche. È necessario allungare gli orari delle prestazioni, assumere più personale, dare formazione e centralità ai medici. Si parla sempre di costi, necessità e difficoltà nel reperire le risorse, ma le risorse del MES sarebbero subito disponibili. Perché il Governo si ostina a non volerle utilizzare? Occorre concentrarsi sulla medicina territoriale: distretti, ambulatori, assistenza domiciliare, gestione della cronicità, vicinanza ai più deboli, residenze socio-sanitarie. Questi fondi tanto bistrattati potrebbero servire a rimodernare tutte quelle apparecchiature vetuste, che costano più di manutenzione che non di utilizzo; tutti quei vecchi mammografi che danno diagnosi sbagliate a pazienti con falsi negativi e poi devono essere operate urgentemente per tumore della mammella. Mettiamo da parte le ideologie e cerchiamo di essere pratici, senza ricorrere ad altri sistemi che porterebbero a creare nel nostro Paese un debito più alto. Se vogliamo imparare una lezione da questo periodo dobbiamo provare a lasciarci alle spalle l'Italia degli ospedali incompiuti e le assunzioni in sanità come bacini elettorali di persone incompetenti. A proposito degli ospedali, mi aspettavo che nel decreto semplificazioni, visto che nello Stato ci sono 6 miliardi destinati all'edilizia sanitaria, si potesse fare qualcosa per sbloccare le pratiche farraginose che le Regioni devono fare per usufruire di questo fondo. Il decreto semplificazioni sarebbe stato l'ideale. Comunque ho visto anche che nel decreto agosto...

anello di congiunzione tra le Regioni e lo Stato. Al di là del fatto che ho visto il numero di assunzioni, per cui si arriverà che ci sarà un dirigente per ogni sei dipendenti (mi sembra un po' troppo, ma si vede che servirà), soprattutto Ministro le chiedo: come mai è stata commissariata l'Agenas? Se è stata commissariata, cosa è cambiato adesso per cui è stato tolto il commissario, cioè non è più commissario, ma è direttore generale? Una persona di specchiata professionalità (quindi nulla da dire), ma mi chiedo solo perché l'Agenas sia stata commissariata in un momento in cui il Paese avrebbe avuto assoluta necessità

Ministro, onorevoli colleghi, noi non possiamo trattare di queste comunicazioni se non inserendole all'interno di tutti i documenti e i provvedimenti che questo Governo sta assumendo. Gli italiani ormai hanno capito che ogni Governo si porta le persone di propria fiducia, quelle che ritiene di maggior competenza, quelle di cui si fida per professionalità. E fin qui è tutto chiaro. ci chiediamo per quale motivo ignoto voi continuiate ad assumere gente nei vari Ministeri se poi scegliete di avvalervi di comitati *ad hoc*. Perché non utilizzate le competenze le competenze dei funzionari presenti all'interno dei Ministeri? Se li avete assunti, evidentemente ve ne era necessità; se continuate ad assumerli, evidentemente vi è ancora necessità. Ma voi, poi, continuate a utilizzare i vostri comitati. Mi comitati. Mi rivolgo anche agli italiani, perché già nel 2018-2019 la Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 del suo Ministero aveva attivato un gruppo di lavoro per approfondire le capacità di fronteggiare eventi con un grande numero di vittime; quel gruppo di lavoro ha prodotto un piano che voi avete messo in un cassetto.

sugli scenari di diffusione del Covid-19 nel caso in cui il virus non potesse essere contenuto localmente, e voi lo avete messo in un cassetto, lo avete secretato. Voi avete scelto consapevolmente e colpevolmente, Ministro, di non fare nulla, con tutte le conseguenze che purtroppo molte famiglie italiane hanno subito, salvo poi continuare a scaricare le responsabilità sulle Regioni - come fate ora - o sui dirigenti scolastici e sugli enti

i casi sono due, Ministro: o non sapete fare programmazione o non la volete fare. Io non so che cosa sia più grave, ma so per certo che tutti gli italiani stanno pagando la vostra Inoltre, se questo Governo si è fatto trovare impreparato di fronte all'epidemia a febbraio, dopo sette mesi dovrebbe essere qui con uno straccio di piano strutturale per affrontare l'emergenza;

quattro mesi? Per quanto tempo, Ministro, volete prorogare quelle misure? Vi è un'improvvisazione continua da parte vostra su tutti i settori e ne sta risentendo la nostra economia, i nostri giovani e l'attrattività del nostro Paese. Ve lo ha detto anche Draghi: dovete cambiare rotta. Oggi lei avrebbe dovuto venire qui a dirci che il Governo era pronto per affrontare una seconda ondata. Evidentemente io sono eccessivamente ottimista, perché questo mi sarebbe sembrato di buon senso, e invece nulla. Lei avrebbe dovuto dirci che cosa fare e come pensate di farlo; lei dovrebbe essere qui a dirci qual è l'idea del futuro per il nostro Paese. A un anno, a tre anni, a cinque anni, quali sono, Ministro, le riforme strutturali che pensate di mettere in atto per

e dopo che cosa fate? Date loro un foglio di via, così vanno a ingrossare le file della malavita, oppure andate a ripristinare il *business* delle cooperative? Quale delle due, Ministro?

che avete chiuso le scuole a febbraio e a meno di dieci giorni dall'inizio siete ancora completamente in alto mare? Gli italiani vedono chiaramente che siete completamente impreparati. Voi state giocando con il futuro degli studenti e con l'amore dei genitori per i propri figli. I nostri ragazzi hanno diritto di andare a scuola: è un diritto costituzionalmente garantito.

a partire dalla prima dichiarazione del Governo che ha decretato lo stato di emergenza nazionale per pandemia da Covid-19 (era il 30 gennaio 2020), il popolo italiano ha reagito a questo tsunami con una maturità che mai ci saremmo aspettati. I nostri medici hanno fatto più del loro dovere, tanto da essere definiti «eroi»; alcuni hanno anche sacrificato la loro vita per curare i pazienti colpiti da questo subdolo virus. I cittadini italiani hanno accettato con disciplina tutte le regole e le misure di contenimento possibili e inimmaginabili; limitazioni notevoli di diritti fondamentali come quello alla libertà di circolazione, di studio, di lavoro e persino alla propria sicurezza: penso - ad esempio - anche alle famiglie costrette a vivere durante il *lockdown* situazioni di violenza domestica. Eppure gli italiani, a differenza di altri popoli europei, si sono dimostrati in tutto questo uniti, compatti, maturi e responsabili, a volte più di qualche rappresentante politico. Accettando tutte queste restrizioni, l'isolamento in casa e persino un forte indebitamento pubblico hanno fatto scendere i contagi da Covid-19 a percentuali bassissime, tra le più basse in tutto il mondo. È indubbio, pertanto, che le politiche attuate in Italia dal Governo al fine di combattere e contenere la pandemia si siano dimostrate estremamente efficaci, e per questo la ringraziamo, signor Ministro. Altrove, invece, a causa dell'incapacità di alcuni governanti, il virus si è diffuso in maniera incontrollata: penso agli Stati Uniti, al Brasile, all'India dove addirittura si sono registrati 80.000 casi in un giorno, ma anche alla Spagna e alla Francia. Ebbene, ora non possiamo vanificare questi risultati; dobbiamo tornare a essere uniti e responsabili; proteggerci e proteggere gli altri è un dovere civico. Dopo la prima e la seconda fase, bene ha fatto il Governo a consentire la ripresa di tutte le attività imprenditoriali dell'economia, del turismo. Purtroppo il virus non è andato in vacanza, ma è venuto con noi, e le misure di contenimento non dovevano essere assolutamente disattese, soprattutto da certe Regioni. I contagi sono ripresi e bene ha fatto lei, signor Ministro, il 16 agosto a ordinare la sospensione delle attività del ballo in luoghi aperti e chiusi, nelle discoteche in altri spazi a ciò adibiti, nonché a imporre l'uso della mascherina nei luoghi a rischio assembramento dalle ore 18 alle ore 6 del mattino. Purtroppo, però, l'esodo dei vacanzieri dalle Regioni interne del Paese alle coste ha fatto dimenticare a tutti che siamo ancora in stato di emergenza sanitaria e che il virus esiste ancora, non è sconfitto, ma è ben presente ed è pronto ad abbatterci di nuovo. È irresponsabile e pericoloso minimizzare i suoi effetti, negarne addirittura l'esistenza o disincentivare l'uso della mascherina, come hanno fatto e continuano a fare qualche politico e qualche imprenditore. In Sardegna, la mia Regione, li chiamiamo prenditori, perché vengono per trarre profitto, approfittando delle nostre bellezze naturali, ma lasciano ben poco agli abitanti dell'isola. Sì, i soldi se li portano via. Quest'anno, prenditori senza scrupoli hanno anteposto il diritto al divertimento e il loro profitto al diritto alla salute dei cittadini. Il risultato è stato quello di una ripresa dei contagi, ma il risultato ancora più grave che ne è scaturito è stato quello di un attacco mediatico alla Regione Sardegna senza precedenti e immotivato,

quello che ritiene. Quando verrà il suo turno, dirà quello che vuole. Prego. Da isola Covid *free* si è passati in un attimo a Regione pericolosa secondo i *media*, ma così non è. Non esiste un caso Sardegna, come ha detto il vice ministro Sileri: esiste una ripresa dei contagi a causa di vacanzieri irresponsabili e imprenditori superficiali e a danno dei sardi che lavorano e si sono impegnati nel settore del turismo e non solo in Costa Smeralda, perché la Sardegna non è la Costa Smeralda. La Sardegna è fatta anche di coste bellissime, incontaminate, e soprattutto delle zone interne. Qualcuno dei nostri rappresentanti politici non riesce ancora a capire che il pericolo Covid non è un pericolo a noi esterno, come possono essere una tromba d'aria, un terremoto, un vulcano in eruzione, per cui per stare lontano da quel pericolo basta non andare nel luogo dove c'è l'evento calamitoso. Il pericolo Covid risiede in ognuno di noi: siamo noi che, senza consapevolezza, magari positivi asintomatici, non utilizzando la mascherina, non rispettando la regola del distanziamento sociale, contagiamo gli altri, i quali a loro volta tornano a casa da padri, madri e nonni contagiandoli. *(Applausi)*. In questa catena qualcuno viene colpito più gravemente di altri e non ce la fa. Ecco che allora il distanziamento sociale e la mascherina diventano fondamentali misure di prevenzione che aiutano a contenere questa catena di contagi. auspico che i cittadini conservino maturità e prudenza; che il Governo sappia misurare aperture e restringimenti; sappia far ripartire questo Paese boccheggiante con investimenti soprattutto nella sanità, nella medicina territoriale, che abbiamo quasi distrutto e che invece oggi stiamo riscoprendo fondamentale. Occorrono solo sempre più urgenti un coordinamento, una strategia comune con gli altri Paesi europei, un Consiglio straordinario di tutti i Ministri della sanità europei. Se vogliamo sconfiggere la pandemia, ogni Stato non può più procedere per conto suo. Chiudere le frontiere - come ha fatto ieri l'Ungheria di Orbàn, Paese che ha avuto contagi bassi per tutta la pandemia, ma che ha fatto pochissimi *test* - non è una soluzione, perché gravissimi sarebbero gli effetti sull'economia di tutta la comunità europea.

Dopo un inizio difficilissimo, in cui l'Italia è stata per alcune settimane l'epicentro mondiale del virus dopo la Cina, il nostro Paese ha saputo affrontare in modo efficace e lungimirante il contenimento del Covid, come ci ha detto nel suo intervento poco fa. È sufficiente osservare i recenti numeri relativi alla diffusione dei contagi in relazione a quelli di molti altri Paesi europei (e non solo) per valutare l'adeguatezza delle soluzioni messe in campo dal Governo con l'indispensabile collaborazione degli scienziati. Attualmente i focolai sono sotto controllo, nonostante l'incremento dei casi legati agli spostamenti estivi, grazie al sistema investigativo dietro il *contact tracing*. È del tutto evidente che la sfida che abbiamo davanti, che si fonda sulla necessità di tenere insieme il diritto alla salute con la salvaguardia del sistema economico e sociale e gli interessi collettivi con quelli individuali, passa dalla nostra capacità di rendere ancora più efficace questo sistema. Rapidità di intervento e abilità di risalire ai casi sospetti attraverso la ricostruzione dei contatti del contagio sono le chiavi della capacità di contenere. Non è un caso che quasi il 32 per cento delle diagnosi con tampone avvenga grazie a quest'attività, come riporta l'ultimo riferimento dell'Istituto superiore di sanità. Oggi sono stati fatti 103.000 tamponi. Per aumentare la nostra capacità di resilienza stiamo aumentando il numero di *test* diagnostici ed è importante che lei, signor Ministro, abbia confermato poco fa questa volontà, questo indirizzo strategico. Infatti, i tamponi sono uno strumento non soltanto di diagnosi, ma anche di sorveglianza attiva. Se è fondamentale che i cittadini rispettino le norme di distanziamento sociale e usino i dispositivi di protezione individuale come le mascherine e l'igiene a cui lei ha fatto riferimento nella sua esposizione - che sono uno strumento fondamentale per impedire il contagio; dall'altra parte la responsabilità dei singoli non è sufficiente senza la capacità dello Stato di procedere a una sorveglianza intensificata della trasmissione nelle nostre comunità. E si tratta di una questione non solo sanitaria, ma anche economica perché non ci può essere vera ripresa senza un controllo dell'epidemia. In questo senso eviteremo i guai che stanno cominciando ad affrontare molti Paesi se sapremo tenere insieme la responsabilità sociale e civica diffusa. Chi rappresenta le istituzioni politiche sta esercitando proprio il dovere etico e civico di prendersi cura della salute e rispettare le regole comuni essenziali che ci siamo dati in questo momento e non dare il cattivo esempio invitando a disobbedire a minime norme di sicurezza, minando l'efficacia delle misure messe in campo per impedire una recrudescenza del contagio. Sto parlando di norme per tutelare la comunità e, soprattutto, i soggetti più fragili. Qui, infatti, si tratta non di difendere la libertà, ma di un deliberato tentativo di mettere in discussione le misure precauzionali e le raccomandazioni con cui il mondo scientifico e le istituzioni stanno cercando di proteggere la salute pubblica e impedire un ulteriore *lockdown*, che metterebbe definitivamente in ginocchio il nostro Paese. Nessuno vuole costringere i cittadini a chiudersi in casa. È vero l'esatto contrario: per essere liberi dobbiamo essere responsabili, perché deve essere chiaro a tutti che il virus è sempre qui e l'unico modo che abbiamo per continuare a vivere la nostra vita è mantenere le precauzioni. Chi racconta il contrario è un irresponsabile che non ha a cuore la tutela della salute pubblica, diritto fondamentale costituzionalmente garantito. A tale proposito non possiamo tacere il nostro dovere di gratitudine nei confronti delle tantissime persone che hanno fronteggiato e stanno ancora fronteggiando il Covid, a partire dal nostro straordinario personale sanitario alla memoria di quelle persone che, a causa della malattia, hanno perso la vita o i loro cari. Non bisogna minimizzare mai i pericoli e i rischi che l'Italia corre ancora oggi, anche se i malati, per fortuna, sono molti di meno e non siamo in emergenza. Vorrei inoltre riconoscere al Governo, per il suo tramite, signor Ministro, l'impegno con cui si è cercato di affrontare la riapertura delle scuole, poiché deve essere chiaro che è una sfida grandissima che riguarda tutti i Paesi. La scuola è la più importante struttura del Paese. E non dimentichiamo che in Germania hanno chiuso più di 100 scuole con 350 insegnanti e 6.000 alunni in quarantena. Il lavoro fatto dal Governo e dalle Regioni darà i suoi frutti solo in un clima di collaborazione tra istituzioni sanitarie, attraverso un serio patto educativo tra docenti, famiglie e studenti, con uno sguardo di attenzione particolare a bambini e ragazzi che, in ragione di alcune patologie e disabilità, dovranno affrontare questo momento non senza paura, e che devono essere costantemente tutelati. Due giorni fa, Ministro, al *summit* dell'OMS Europa ha sottolineato proprio l'importanza di farci trovare pronti in caso di chiusure temporanee, perché lo stop della didattica può provocare effetti gravi in termini di istruzione e di salute, compresa quella emotiva, sullo sviluppo sociale e con il rischio di trovarsi in un ambiente familiare violento. L'impatto è pesante, ancor più per i bambini in situazioni vulnerabili e di indigenza e perciò bisogna fare in modo che tutti continuino ad avere accesso agli apprendimenti, anche in situazioni di emergenza. Allo stesso modo sarà importante continuare a garantire - nel caso di una recrudescenza del virus - i servizi alle persone più fragili con disabilità, agli anziani che, più degli altri, hanno sofferto nel *lockdown* nella fase iniziale.

automaticamente)...* considerato che la maggior parte di loro ha qui l'unica possibilità di relazione esterna alla famiglia. ci aspettano mesi difficili, ma li stiamo affrontando con la giusta consapevolezza politica, etica e sociale; la stessa che ci ha spinto ad essere prudenti nei mesi scorsi. Il quadro potrebbe mutare da un momento all'altro, ma ora abbiamo gli strumenti per affrontare i cambiamenti. Il Paese ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, ma anche sociali ed economici, ma la salute dei cittadini viene prima di tutto il resto, e il virus, combattuto in tempi più rapidi che altrove, deve continuare a essere contrastato. Adesso sta ad ognuno di noi vivere la normalità conquistata in sicurezza, rispettando le regole per fare... Per cortesia, concluda davvero. IORI *(PD)*. ... oltreché anche l'economia appena ripartita non si fermi. Sono certa che continueremo a essere prudenti tenendo a mente la terribile lezione dei mesi scorsi. Serve ancora continuare a rispettare noi stessi e gli altri in un incessante lavoro di cura di sé e dell'altro, che è l'unica strada per tenere in piedi il nostro Paese.

accogliamo sempre con molto piacere in quest'Aula per il suo garbo istituzionale, che non è cosa frequente nei membri del Governo e comunque della maggioranza e della politica in genere. Lei invece ha da sempre un tratto distintivo e dice le cose che ci fa piacere sentire e quelle che non ci fa piacere sentire, ma mantenendo sempre un garbo istituzionale, che non è così diffuso; e ciò, naturalmente, ostacola anche i rapporti tra opposizione e maggioranza, perché con una

nel corso dei quali l'attività normativa e regolamentare del Governo è stata abbastanza altalenante e vorrei dire - usando un termine medico - qualche volta anche schizofrenica. 16 decreti-legge, con disposizioni più volte integrate e modificate, che prevedono circa 300 provvedimenti attuativi; 16 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 6 delibere del Consiglio dei ministri; 40 ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; 11 ordinanze del commissario straordinario; 17 decreti o comunicati dei diversi Ministeri coinvolti nella pandemia; 72 provvedimenti della Protezione civile. Questa è una delle ragioni per cui si era chiesto un intervento più ampio in quest'Assemblea, da parte del presidente Conte, che riguardasse sicuramente i temi attuali della sanità, ma che coinvolgesse anche i temi dell'economia della ripresa economica, laddove dovesse esserci ed essere più evidente, e anche i dati drammatici che ci propina periodicamente l'INPS sull'occupazione. Questo è il motivo per cui, senza nulla togliere a lei, signor Ministro, avremmo gradito avere un'interlocuzione più ampia sullo stato attuale del nostro Paese, in questo momento. Per quanto riguarda lei, su ciò che ha detto, signor Ministro, credo di non avere nulla da ridire: ha fatto uno spaccato della situazione, partendo dal livello internazionale, da ciò che si sta facendo a livello mondiale, per passare al livello europeo e poi determinare i passi da fare nella nostra Nazione, per evitare una recrudescenza o un ritorno del virus; virus; quei passi che già dall'inizio avevate dichiarato, e cioè il distanziamento sociale e il *lockdown*, che hanno avuto sicuramente un effetto ampiamente positivo,

Su questo ritengo che non ci sia veramente nulla da dire. Quello che invece mi preoccupa, signor Ministro, è quello che lei non ha detto: non ha parlato delle criticità attuali del nostro sistema sanitario,

stancanti e affaticanti. E questo lo può dire una persona che ha un'esperienza diretta in tale settore.

alla grandissima difficoltà per ridurre le liste d'attesa, signor Ministro. Le liste d'attesa non si stanno per niente riducendo, ma si stanno allungando. questo è dovuto al fatto che mentre prima, per effettuare una visita, bastava entrare in un ambulatorio o in un poliambulatorio

Di ciò avrei voluto sentir parlare: come della questione di ridurre i tempi di attesa, che sono veramente molto lunghi e preoccupanti per tutta la categoria sanitaria.

termini di sanità. In questo periodo di pandemia, soprattutto nella stagione estiva, la Sardegna ha avuto un sovraccarico; ci fa piacere che questo sia avvenuto e avremmo voluto ancora adesso avere tantissimi turisti.

per un accordo Stato-Regione, ci sono sistemi compensativi diversi dalle altre Regioni. Ponga però attenzione, perché il sistema anche in Sardegna ha necessità di un intervento veramente forte e importante. avremmo voluto proseguire con l'attività turistica; io sono uno di quelli che ringraziano i turisti, perché vengono a trascorrere - penso sempre con piacere - le loro vacanze nella nostra Regione, e non sono tra coloro che rifiutano questo sistema di approvvigionamento economico della Regione. *(Applausi)*. È una voce importante nella nostra Regione, vale quasi il 10 per cento del PIL; si potrebbe fare molto di più e abbiamo subito sicuramente una crisi. Io ringrazio - come ha fatto lei - tutti gli operatori della sanità, tutti indistintamente per la loro prestazione. Ma devo anche ringraziare gli operatori

Presidente, colleghi, il Governo e la maggioranza hanno voluto fortemente la proroga dello stato di emergenza per Lo hanno fatto per tutelare la salute degli italiani o per prorogare i poteri speciali del Governo e del presidente Conte? L'avvocato del popolo ha mobilitato tutto l'Esercito per limitare i nostri movimenti.

alla vera tutela della salute, allora come mai si stanno autorizzando sbarchi e l'entrata di immigrati senza i necessari controlli? Come mai sono lasciati liberi di scorrazzare ovunque con la possibilità di diffondere ancora il virus? Vergogna! Il Presidente della Regione Siciliana si è visto, infatti, costretto a bloccare le entrate per tutelare i suoi cittadini e la risposta del Governo è stata l'impugnativa dell'ordinanza. La cronaca di tutti i giorni narra di centri di accoglienza sfasciati dai nuovi arrivati perché vogliono evadere dalla quarantena. Fanno danni enormi e feriscono i nostri agenti, ai quali non è consentito di difendersi adeguatamente. Non volete dotarli nemmeno del *taser*. Ogni giorno subiscono ferimenti e contagi. Tutto ciò accade contro il popolo italiano, che soffre una disoccupazione dilagante e spesso le famiglie non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena dei loro figli. Poiché non c'è lavoro per gli italiani, anche i nuovi arrivati non avranno occupazione, ma al Governo non interessa nulla e ci costringe a mantenerli di tutto punto, comprese le paghette e quant'altro. Di fatto, ci rende schiavi dei nuovi arrivati. Non parliamo dei reati e dei danni di costoro. Se qualcuno li denuncia, dobbiamo accollarci pure le spese dei loro difensori fino al terzo grado di giudizio. Sono state noleggiate molte navi per la quarantena in crociera e tutto ciò genera costi proibitivi per un Paese come l'Italia con un PIL in caduta libera. (*Applausi*). Visto il benvenuto con il quale riceviamo tutti questi immigrati, i trafficanti di carne umana si stanno già organizzando con capienti barconi per invaderci definitivamente. State favorendo l'epidemia con l'immigrazione di massa. Siete criminali e traditori del popolo italiano. L'*hotspot* di Lampedusa può ospitare solo 192 immigrati e ogni giorno sono sopra il migliaio. Come si vede, le regole del distanziamento valgono solo per gli italiani: vergogna! Non avete freni inibitori nel permettere a cooperative di arricchirsi sulle spalle degli italiani. Ci sentiamo mortificati davanti al mondo per essere governati da democratici rossi, tutti antifascisti DOC, che, contro la volontà del popolo, vogliono imporre l'immigrazione di massa. Il Governo ha voluto la proroga dello stato d'emergenza, ma ancora non ci ha risposto su cosa sta facendo per tutelare la salute degli italiani. Di certo importa positivi a iosa e del semplice vaccino antinfluenzale - e siamo a settembre - non si sa ancora nulla. Il vostro comportamento dissennato e il prolungamento dello stato d'emergenza hanno dato un ulteriore colpo al turismo e un ultimo calcio all'economia nazionale. Come faremo a pagare le ingenti spese che ci costringete a sostenere? Pensate forse al MES sanitario per "incaprettare" definitivamente l'Italia e il suo futuro? Qui siamo in un mondo alla rovescia, dove neanche la fervida fantasia di Orwell era arrivata: chi è pagato per fare gli interessi del popolo italiano fa l'esatto contrario e un Governo tradisce volutamente i suoi cittadini e favorisce altri Stati. È da fine gennaio che è stata decretata l'emergenza per i virus della Cina e ora spunta una relazione del 12 febbraio, prima che in Italia si registrassero casi di coronavirus, con cui gli esperti anticipavano esattamente ciò che sarebbe successo, compresi i 35.000 morti. Sapevano tutto e già a gennaio il direttore generale della programmazione del Ministero della salute parlava di un piano d'emergenza con diversi scenari. Sì, il Governo sapeva, ma ha fatto finta di niente; a Palazzo Chigi, però, non si sono fatti trovare impreparati, si sono dotati di tutto... Non si sono fatti trovare impreparati, si sono dotati di tutto l'occorrente possibile e immaginabile, dalle mascherine ai respiratori con le bombole d'ossigeno. Penso ai molti Paesi esteri che hanno chiesto conto alla Cina della pandemia che ha provocato. Qui da noi, il silenzio più assoluto, neanche una parola. I giorni scorsi un Ministro cinese ci ha fatto nuovamente visita. Come mai questo interesse e questi contatti con il nostro Governo? Forse perché la bandiera cinese ha cinque stelle, come quella dei 5 Stelle nostrani? In conclusione, fino a quando dobbiamo tollerare una situazione simile? Non ne possiamo più di comportamenti contro gli italiani. Signor Presidente Mattarella, per favore, intervenga: mandi a casa questo Governo.

in quest'Aula si può discutere di tutto e, come lei dice, spesso ognuno ha le sue opinioni e siamo tutti in ascolto di quello che dicono gli altri in maniera rispettosa. Credo però che sentirsi dare dei "criminali" sia una cosa grave e non lo posso accettare.

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per il nostro Paese, a tratti drammatici. Le circostanze ci hanno messo di fronte a scelte difficili. Abbiamo dovuto operare in scenari inediti all'inizio di una pandemia che poi, via via, purtroppo ha colpito tutto il mondo. Il Governo ha saputo prendere le decisioni più appropriate, agendo con tempestività e risolutezza e tutelando la salute e gli interessi pubblici. Questo *modus operandi* è stato preso da esempio da altri Paesi, che dopo di noi sono stati colpiti, purtroppo, dalla pandemia. Lei, signor Ministro, ha giustamente sottolineato il comportamento degli italiani che durante le settimane del *lockdown* sono stati ligi alle regole e in questo modo hanno consentito di far diminuire in poco tempo la curva dei contagi, che ad un certo punto sembrava difficilmente arrestabile. È stato un successo del Paese, non di questa maggioranza o di questo Governo, come lei ha precisato. È un successo degli italiani e in particolare degli operatori del comparto sanitario, che hanno lavorato senza sosta, prestandosi a turni massacranti spesso sopperendo, con la loro abnegazione e il loro senso del dovere, alle carenze di un sistema sanitario nazionale che era stato depauperato nel corso degli ultimi decenni. degli ultimi decenni. Tengo molto a sottolineare che l'urto della pandemia è stato retto dalla sanità pubblica. Questi sacrifici sono stati fondamentali e ciò è tanto

hanno salvato dalla morte 3,2 milioni di persone. In Italia le morti evitate, secondo questo studio, sono state 630.000. Di sicuro ci sarà chi non crederà a tali risultati e allora magari potrà guardare non a uno studio predittivo come questo, ma quello che di terribile è successo nei Paesi che hanno fatto una scelta diversa dalla nostra. Cito ad esempio il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile e molti altri

i loro Paesi dopo il nostro e quindi avessero un precedente su cui basarsi per adottare i provvedimenti più opportuni per contrastare il dilagare del contagio. I numeri mondiali della pandemia che lei ha citato, signor Ministro, dimostrano che in questa vicenda non c'è nulla nulla di ideologico: non c'è destra né sinistra; non c'è chi è coraggioso e sfida il contagio o chi è fifone e si protegge. In gioco ci sono solo ed esclusivamente la salute di miliardi di persone e il loro diritto a essere protetti dal contagio, adottando tutte le buone pratiche approvate dalla comunità scientifica internazionale. Di fronte a queste evidenze, ai morti, alle bare trasportate dai camion militari, c'è ancora chi sostiene che sia tutto un *bluff*

Stamane, quindi non solo pochi minuti fa, c'era ancora chi parlava di dittatura sanitaria in atto in Italia. Altri negazionisti, qualche settimana fa, hanno organizzato un convegno in questo edificio, rifiutando di indossare la mascherina e invocando la libertà personale, salvo poi essere indirettamente redarguiti, qualche ora dopo, dal Presidente della Repubblica che, dall'alto della sua autorevolezza, ha giustamente precisato che nessuno ha la libertà di far ammalare altre persone. Quella non è libertà, ma ignoranza, menefreghismo, cinismo e incoscienza: quello, e non altro. *(Applausi)*. Il partito dei negazionisti non accenna a sgonfiarsi, anzi forse si ingrossa e tra le sue fila entra non solo chi ignora il pericolo o lo sottovaluta, magari in buona fede, per pura ignoranza, ma soprattutto vi entra direi a pieno titolo - chi mira ad avere notorietà mediatica o voglia spuntare uno zero virgola in più nei sondaggi elettorali. Ciò detto, le azioni da mettere in pratica nell'immediato futuro sono note e passo velocemente a elencarle: dobbiamo proseguire sulla strada della massima attenzione, della prudenza e della salvaguardia della salute pubblica e si dovranno potenziare tutti gli strumenti che consentono d'individuare con tempestività l'insorgere di nuovi focolai, così da poterli circoscrivere immediatamente. Di conseguenza, sarà necessario potenziare sia gli strumenti per la diagnosi, sia le strutture che possono eseguirla, anche superando i localismi regionali, che a volte hanno generato una pluralità di iniziative che poi si sono rivelate controproducenti. Signor Ministro, lei poc'anzi ha citato la necessità di adottare misure di reciprocità con gli altri Paesi, facendo per esempio test negli aeroporti sia per chi entra nel nostro Paese, sia per gli italiani che escono dal territorio nazionale. L'obiettivo dev'essere quello di ritornare al più presto alla normalità e quindi consentire la ripresa di tutte le attività economiche e sociali in totale sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia in ambito nazionale e internazionale. L'anno scolastico riprenderà, com'è stato già deciso, con le lezioni in presenza, adottando tutti gli accorgimenti per assicurare la salute dei nostri studenti, ad esempio norme banali, ma utilissime, come il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale di un metro e, ove ciò non fosse fisicamente possibile, utilizzando le mascherine. Nelle sue comunicazioni, signor Ministro, ha sottolineato l'esigenza di riavvicinare la scuola al Servizio sanitario nazionale, costruendo una sua relazione organica organica con le aziende sanitarie territoriali che non lasceranno soli, come ha ripetutamente detto, le scuole, gli studenti, i presidi e i docenti.

Infine, grande attenzione dovrà porsi sul trasporto pubblico e, in particolare, su quello scolastico dedicato, le cui linee guida sono state pure recentemente approvate in sede di Conferenza unificata ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze la fruizione di tali servizi in condizioni di piena sicurezza. Come si vede, non siamo "criminali", ma operiamo nell'esclusivo interesse degli italiani. *(Applausi)*.

ringrazio di avermi dato la parola. Non so perché tocchi a me parlare per primo, ma lo faccio volentieri, per dire che ho ascoltato con attenzione il Ministro e le sue parole garbate. Lei, signor Ministro, è una delle poche persone al Governo che, se non altro, esprime le proprie idee, magari assai diverse dalle mie,

ci riconferma che la nostra speranza sta nelle tre regole essenziali: le mascherine, la distanza e la pulizia personale; *grosso modo*, tranne le mascherine, è ciò che una buona educazione, già da qualche secolo, dovrebbe insegnare ai giovani. Poi, al di là di queste regole di buon comportamento,

sulla possibilità che si arrivi a un vaccino e sul fatto che adesso forse cominciano corsi di formazione. Dopo le speranze, ci fa qualche promessa: ci dice che non lasceremo soli i presidi (che stanno tremando, perché non lasciarli soli va bene, ma bisogna vedere che vicinanza darete

Poi ci dice, sempre lei - l'ho ascoltata con attenzione, garbatamente - che la nostra priorità oggi è la riapertura delle scuole. Mi chiedo, signor Ministro,

Allora, se questa è la vostra priorità, mi sento male: figurarsi quelle che non lo sono! *(Applausi)*. Se la vostra priorità porta alla necessità di far intervenire le Forze armate le Forze armate! - per sostituire i bidelli nel consegnare i tavolini (immagino che i bidelli li manderemo a controllare i centri di prima accoglienza, perché non scappino gli immigrati, così sarà completa la costruzione di questo Governo), male mi sento. Per voi la scuola è la priorità e oggi i genitori non sanno che fine faranno i loro figli, come mangeranno nelle mense scolastiche, se potranno andare con gli autobus, in quanti e come e se potranno portare o meno le mascherine in aula.

Pellegrini

che il 6 febbraio di quest'anno uno studio diceva: state attenti, possono esserci 60.000 morti. E fino al 21 febbraio, però - solo perché è arrivato il primo caso - il Governo non ha fatto niente; anzi, andava andava a fare aperitivi per dire che non c'era problema. Allora, è eccessiva la libertà che questo Governo, negazionista, ha

vorremmo la trasparenza sull'oggi. Continuo a leggere su tutti i giornali le statistiche della malattia. Tenga presente che non sono negazionista; tutt'altro: ai miei figli dico di stare attenti, di non frequentare luoghi troppo affollati e di usare le mascherine. Voglio capire bene, però: perché le statistiche che ci date date sono così negazioniste della capacità di comprensione? Perché non ci dite chi è veramente malato e chi è contagiato senza essere malato? Perché non ci dite il numero di coloro che sono contagiati senza essere malati, cioè gli asintomatici, che a loro volta possono forse contagiare, certamente contagiare o sicuramente non contagiare?

Ci volete dare un'informazione corretta? Io la tengo la mascherina, allora, consapevole però che il mio rischio di andare in terapia intensiva è quello di 107 italiani su 50 milioni; non devo terrorizzare l'Italia non devo terrorizzare l'Italia facendo credere che da un momento all'altro milioni di persone possano finire in terapia intensiva. Chiediamo un protocollo immediato per la scuola: oggi lo vogliamo e lo volevamo ieri. Chiediamo la verità, signor Ministro, sull'emergenza immigrazione. Non si può essere allarmisti su tutto, tranne che su un caso conclamato di pericolo di contagio, e non perché siano di un altro Continente, perché lì il controllo sulla malattia è arrivato dopo e male. È quindi evidente che da lì proviene un rischio: c'è per i Paesi stranieri in genere e lì ancora di più. E se questi soggetti scappano appena arrivano? Quando parliamo di blocco navale, oddio di cosa parliamo! Il blocco degli italiani nelle case è possibile - è stato giusto, quando c'è stato, ma lo si paventa ora che è inutile - ma quello degli immigrati fuori dal nostro territorio diventa una bestemmia. Com'è possibile? Allora c'è un dato ideologico ed evidentemente di convenienza nell'affrontare il tema del contagio. Vorrei che, come ci ha chiesto, fossimo davvero tutti sulla stessa barca

ha concesso. Siamo assolutamente convinti che bisogna affrontare davvero insieme quest'evenienza, sia quando occorre massima severità, sia adesso, in un momento in cui non è più assolutamente nella del Governo fare tutto da solo secondo i propri usi, le proprie convenienze e le proprie non accettabili priorità. *(Applausi)*.

diffuso e le famiglie italiane in queste ore e in questi giorni stanno discutendo di come possono organizzarsi, di come la scuola ripartirà e del fatto che, ad esempio, probabilmente non potranno più avere l'aiuto e il supporto dei nonni, per timore che i ragazzi e i bambini possano contagiarli. È questo che stanno vivendo le famiglie italiane e dobbiamo essere loro vicini.

lo è la questione della famiglia allargata, grazie ai nonni che aiutano con i bambini. Questo stiamo vivendo. Sono particolarmente contenta, signor Ministro, che abbia ricordato il dibattito che abbiamo fatto il 10 agosto in

La prima è quella che ha ricordato, che ha preso provvedimenti sui tamponi da fare ai nostri concittadini che erano andati in Croazia, Spagna, Grecia e Malta: lo si sta facendo sempre di più e si è fatto ogni giorno. Ha ringraziato più volte il personale sanitario e anche in questa fase dobbiamo ringraziare il personale che sta realizzando i tamponi nei porti, negli aeroporti nei *drive-in*; se c'era qualcuno che aveva diritto di fare le ferie in questo periodo era il personale sanitario, che è stato fortemente preso da un lavoro immane, ma molti hanno dovuto interrompere le proprie ferie per essere presenti sul posto di lavoro e realizzare tamponi e test ai nostri concittadini che sono rientrati dalle ferie trascorse in questi Paesi. Penso che quest'ennesima esperienza debba farci capire che non possiamo più trovarci nella condizione di non attivare subito efficaci e immediati tamponi sui nostri concittadini che

arrivare a una comunità europea che non si disturbi per i tamponi reciproci tra Paesi, che devono essere invece all'ordine del giorno, perché l'epidemia si combatte insieme.

ma alcune Regioni hanno derogato alla normativa nazionale che ha ricordato, consentendo la riapertura delle discoteche. Penso che tutta l'Italia debba riflettere su questo punto.

fare tesoro di questa brutta esperienza. Sono convinta che dobbiamo fare appello, come ha fatto più volte, al senso di

però dobbiamo riflettere su questo punto, su cui tornerò infine. Bene, quindi, il tracciamento che stiamo realizzando. Ho sentito, anche

Penso che questa sia l'unica arma che abbiamo per isolare e tracciare l'epidemia, soprattutto in vista dell'inizio dell'attività

penso che dovremmo mettere i termoscanner nelle scuole, per avere un unico sistema di misurazione della febbre, perché è complicato dare alle famiglie anche la responsabilità di misurare la febbre a casa.

previsti: quello all'istruzione e quello alla salute. In questi mesi difficili abbiamo molto parlato di un necessario equilibrio tra libertà individuale e restrizione di tale libertà.

è quella di rafforzare il sistema sanitario, attraverso lo sviluppo della medicina territoriale e di quella scolastica; il Ministro l'ha ribadito anche adesso. Quindi, signor

intendo evitare ogni polemica e vorrei proporre un ragionamento anche ai colleghi dell'opposizione, fermo restando che tutte le critiche e le accuse al Governo nella dialettica politica sono legittime, quando non sono strumentali e false. A mio parere, dovremmo quantomeno provare a metterci d'accordo su alcuni punti fondamentali, che non negano in alcun modo la dialettica tra le diverse posizioni. Il primo: il *lockdown*, che ha prodotto e portato con sé tanti problemi - penso all'economia, ovviamente - comunque ha funzionato, e credo sia un valore per tutto il Paese riconoscere, come ha fatto il Ministro, il risultato non di una parte, tantomeno del Governo o delle Regioni, ma di una comunità. Spesso in Italia accade che nei momenti più difficili la comunità riesce a trovare la capacità di stare insieme e di rispondere anche oltre, e a volte meglio, delle sue classi dirigenti; nella storia, questo è capitato diverse volte. Ciò ci dovrebbe consentire, colleghi, di evitare

Perché dobbiamo cercare di trovare un secondo punto che ci potrebbe unire e qual è questo secondo punto?

Non scherzerei sul tema del negazionismo, perché vorrei fosse chiaro il problema non è legato alla dialettica in queste Aule. Quando in un Paese come la Germania vediamo marciare 10.000 persone che negano il Covid,

che non dovremmo prendere alla leggera e che riguarda il tema del rapporto tra la libertà - la mia libertà la qualità e la sicurezza della mia comunità e il modo in cui siamo in grado di sintetizzarlo, a prescindere dalle diverse posizioni politiche. è arrivato il momento di fare questa discussione, senza gettarci la clava gli uni contro gli altri, ma cercando una via, che ci proponga una sintesi.

Lo dico non per fare delle critiche e con grandissimo rispetto della scienza, ma ad un certo punto una sintesi sulle mascherine, sul metro dinamico e sul metro statico,

la continua discussione dialettica, in cui ad un certo punto si perde il filo.

pesa di più un dato rispetto ad un altro. Guardate che questo aspetto è decisivo per la ripresa economica e voglio dirlo: ne sono convinto fin dall'inizio. La crisi economica è pesantissima e drammatica, ma se vogliamo dare certezza alla ripresa, dobbiamo avere risposte scientifiche certe e dobbiamo essere capaci di portare avanti Quindi, forse è questa la discussione che noi in Parlamento dovremmo fare; potremmo dialogare con il Governo per fare insieme un passo in avanti, senza negare

Siamo prima di tutto noi rappresentanti del popolo a essere più indietro del popolo; non so se mi spiego. Un ultimo punto e ho concluso, signor Presidente. Ministro, sta giustamente lavorando ad un piano. Da questo punto di vista io sono d'accordo con i colleghi dell'opposizione che lo hanno proposto: c'è bisogno di un piano strategico per la sanità, dico), collegato agli investimenti, alle necessità e perfino alla discussione sul MES. Un piano puntuale cambierebbe di tono, perché andremmo a parlare del merito e non di posizioni astratte o ideologiche. Ma questo piano, signor Ministro, deve

e invece non stiamo costruendo il ponte tra il territorio e l'ospedale, tra l'alta competenza e la diffusione Forse è arrivato il momento di porsi l'interrogativo se dobbiamo riportare le RSA nel sistema sanitario nazionale. La mia risposta è chiaramente e nettamente sì, ciò richiede una riorganizzazione territoriale. Sono questi i nodi su cui noi possiamo trovare, cari colleghi, una capacità propositiva del Parlamento. Ripropongo questa idea: facciamo un momento di riflessione in Aula, organizzato strutturato, fondato su competenze scientifiche che ci consentano di dare un contributo e di essere più avanti del senso comune, del discorso del bar, del *tweet*.

ai morti, ma al futuro di questo Paese, quando noi potremo riposarci, ma ci chiederanno perché e che cosa abbiamo fatto ora.

Signor Presidente, ringrazio non ipocritamente il ministro Speranza, perché, essendo Ministro della salute e da un lato sarebbe doveroso per lui, dall'altro, in occasioni più importanti, non toccherebbe solo a lui metterci la faccia, come si suol dire. Il suo tono, come tutti hanno sottolineato, è stato

l'attuale maggioranza o presunta tale non si possa riconoscere, ma ci sono anche cose di buonsenso e, a volte, anche le risoluzioni si valutano per parti separate. Forse poteva avere un po' più di garbo e, invece, ha smentito la pacatezza nell'esprimere

molto controversa e confusa - il tema della scuola è stato dominante; non c'è solo il tema sanitario in senso stretto, ma ci sono anche le ricadute sanitarie su altri aspetti, pensavamo che fosse il Presidente del Consiglio a dover riferire

quelli del MES se senza condizioni e se destinati alla sanità. Lei oggi ci ha detto che bisogna lavarsi le mani e tenere la mascherina. Lo sappiamo e Conte ha preso alla lettera il suo consiglio perché se n'è lavato le mani, ma come fece Pilato: si è lavato le mani. Noi ricordiamo tutti - io sono anche un credente - e abbiamo letto i Testi sacri in cui si parla di Pilato e di quando si lavò le mani. Anche Conte si è lavato le mani e ha mandato Speranza. Non era questa forse l'indicazione che lei dava.

Non saranno decisivi, però il diritto di voto non si valuta sul piano quantitativo. Ogni voto può essere importante. Per quanto riguarda poi le recenti figuracce del Governo potremmo fare un elenco molto lungo, dalla storia dei congiunti, rispolverata per i ragazzi della stessa classe. È stato seriamente detto che sugli autobus quelli della stessa classe potevano stare insieme; adesso si è detto che possono stare insieme se il viaggio dura quindici

voi che state salendo sull'autobus siete nella stessa classe? O doveva memorizzare gli studenti? Forse in un paese piccolo l'autista della corriera lo potrebbe anche fare, ma a Roma, Milano e a Napoli il conducente dell'autobus cosa ne sa se i ragazzi che salgono sono moralmente e tecnicamente congiunti. Avete detto anche cose di questo tipo. Non sappiamo ancora chi deve misurare la febbre. Ministro, poco fa c'era un funzionario dell'università di Tor Vergata che mi diceva che per i test universitari in corso è stato detto prima che bisognava prendere la temperatura nel

non siamo dei sessisti perché l'abbiamo detto anche di Toninelli. Se uno è incapace, lo è indipendentemente dal sesso e il Ministro dell'istruzione non è adeguata a gestire questa fase. Purtroppo, anche chi si occupa di trasporti ha parlato di questa storia

che in Libia ci sono i libici e che i libanesi stanno in Libano. Forse per questo è andato anche Di Stefano con Di Maio in Libia. (*Applausi*). Poi ci sono due Tripoli, ma questo glielo spiegherò un'altra volta a Di Stefano: ce n'è una in Libia e una anche in Libano. Forse da lì nasceva la confusione. Noi siamo assolutamente esterrefatti di di fronte a ciò che ha fatto questo Governo. C'è anche il *caos* immigrazione. Oggi hanno mandato la nave ospedale Allegra perché arriva la Sea Watch. Noi non condividiamo - forse questa è la parte della mozione che a lei non piaceva questa gente e di questi grandi artisti - ho letto che ce n'è uno che ha preso le navi - che sostengono il ritorno della Sea Watch e che incoraggiano il traffico di persone che parte dal Nordafrica. Favoriscono l'arricchimento dei trafficanti. E noi siamo costretti a organizzare la quarantena con le navi, che costa un sacco di soldi. Noi siamo solidali con i cittadini di Lampedusa e con il presidente della Regione Musumeci *(Applausi)* che solo oggi è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio. Forse per questo non è venuto. Speriamo che faccia delle cose buone e che dia delle risposte, anche se dubitiamo che ci saranno. Stiamo riempiendo quindi la Sicilia di navi per la quarantena, stanno arrivando la Sea Watch, Carola Rackete e molti altri. Noi non ci stiamo a tutto questo ed è una politica vergognosa e di resa. Abbiamo dato 11 milioni alla Tunisia giorni fa e gli sbarchi continuano. - guardate un po' - l'autostrada che voleva fare Berlusconi. Ecco, se dovete dire una cosa utile, dovete ridire le cose che hanno detto i Governi di centro-destra, che anche nel Nordafrica hanno fatto una politica di sicurezza e di cooperazione, non di nullità

ci ha detto oggi che saranno resi noti tutti i verbali. Condivido quello che hanno detto molti e che dice anche la nostra proposta di risoluzione.

il 12 febbraio del 2020. Sapevate che cosa avete fatto. Avete anche disatteso le indicazioni delle Regioni. I giornali quest'estate hanno riportato «Blindare Alzano e Nembro» ma Conte ignorò gli scienziati; hanno parlato degli errori e dei ritardi nella settimana di marzo, del giallo delle carte a Conte. E ancora: «Ha mentito pure al Parlamento, il 26 marzo alle Camere il *Premier*

a dire perché ha negato l'evidenza. Ha detto e ammesso addirittura che non aveva letto il rapporto che gli era stato dato i primi di marzo. Ma come? Il Presidente del Consiglio, tutta la discussione che vi è stata? Mandavate alla Cina, di cui siete ormai i camerieri, le mascherine e quant'altro, quando sapevate dell'emergenza

Tenete nascosto tutto. I prìncipi dell'occultismo, siete i negazionisti della verità. Dove è lo *streaming*? Dove è la trasparenza? Dove è il principio "uno vale uno"? Avete occultato documenti e prove per difendere la credibilità di un Governo che è assolutamente inadeguato. Questo ha fatto Conte. Poi può arrivare anche Orano e l'altro pubblico ministero a dire che non ci sono stati i reati. Io spero che invece la procura di Bergamo vada avanti,

riguarda il negazionismo, quelli che fanno i cortei negazionisti sono degli imbecilli. Non ho difficoltà a dirlo perché tali sono. State attenti però perché anche Zingaretti girava sui Navigli a Milano a fare il principe dei negazionisti, anche il sindaco di Bergamo Gori diceva «lasciateci lavorare». Quindi noi non condividiamo la gara al negazionismo, ma non condividiamo neanche l'allarmismo totale. Riteniamo che un clima di emergenza permanente serva solo alla vostra autodifesa politica, alla eternazione del vostro potere. I numeri attuali sono da non sottovalutare, ma siamo a 107 persone in terapia intensiva e i contagiati sono quasi tutti asintomatici. Non dobbiamo sottovalutare nulla, ma l'emergenza permanente non va bene. Non diciamo, quindi, certamente che hanno ragione i negazionisti - che biasimiamo perché non si può giocare con queste cose - ma vorremmo quella trasparenza che non può essere rinviata, Ministro. La trasparenza serve ora e subito, sennò è un'autodifesa per tutti gli errori che avete fatto il 12 febbraio e i primi di marzo,

signor Ministro, come è stato detto in precedenza anche dai colleghi, lei è la vittima sacrificale di questo Governo oggi, di un presidente Conte che abbiamo visto in tutte le trasmissioni televisive durante il periodo di *lockdown*, quando c'era da illudere gli italiani, ma adesso che si arriva alla alla resa dei conti, all'autunno, sparisce e si scioglie come neve al sole. purtroppo il presidente Conte le ha dato il compitino, come al solito. Ricordiamo infatti tutte le volte che il presidente Conte è venuto in quest'Aula: ci diceva «faremo» e «diremo», usava sempre il futuro.

un po' pochino, Ministro, da parte di chi, in questo momento, dovrebbe venire in Senato a spiegare come affronterete l'autunno. Nulla sulle tracciature, nulla sulla distinzione tra contagiato e malato, nulla sulla distinzione tra sintomatico e asintomatico, nulla sulla distinzione tra carica virale Ci viene a raccontare, Ministro, che siamo tutti sulla stessa barca. Ma siete voi sulla stessa barca perché io non voglio essere sulla vostra barca! *(Applausi)*. Noi non vogliamo essere sulla vostra barca perché per mesi,

Il 31 gennaio Conte decreta lo stato di emergenza in assoluta segretezza, senza farlo sapere praticamente a nessuno. Il 7 marzo, Ministro, il Comitato scientifico chiedeva misure rigorose solo in alcuni territori

prendendovi la responsabilità, decidete la chiusura totale di tutta Italia, lo stop agli spostamenti, la chiusura delle scuole e il blocco delle manifestazioni sportive. Vi dovete prendere la responsabilità di quello che avete fatto e non coinvolgerci nella vostra barca che sta affondando. Il 28 marzo arriviamo invece al *cabaret*. Il presidente Conte dice: nessuno resterà indietro, interverremo con misure straordinarie per rilanciare l'economia in modo che l'Italia possa tornare più forte di prima.

L'Istat ci dice, il 7 di luglio, che stima il 38,8 per cento delle imprese italiane a rischio chiusura, lasciando a casa circa 3,6 milioni di addetti,

cento delle aziende dello sport, della cultura e dell'intrattenimento, con circa 700.000 addetti, sono a rischio. Ma non avevate detto che nessuno doveva rimanere indietro? Non l'avevate promesso agli italiani? *(Applausi)*. Non facevate le dirette televisive tutti i sabato sera per far vedere il nostro eroe, presidente Conte, che avrebbe salvato le aziende e le famiglie italiane? E adesso dov'è il presidente Conte? Dov'è? È nascosto? Senza parlare della cassa integrazione: migliaia di italiani stanno aspettando ancora la cassa integrazione. Ma voi con cosa pensate che mangino le famiglie italiane? Col *bonus* vacanza di Franceschini? A proposito di *bonus* vacanza, 2,2 miliardi buttati via; sono stati messi sul tavolo e ne sono stati utilizzati solamente 200 milioni.

accade in un Paese dove prima il 31 gennaio e poi inspiegabilmente il 29 luglio vengono dati pieni poteri al *Premier*, estromettendo il Parlamento dai poteri decisionali. Noi siamo solamente i ratificatori di quello che decide il presidente Conte. Noi dobbiamo semplicemente, secondo voi, dire di sì, perché tutte le volte che diciamo di no non siamo collaborativi, siamo cattivi e non vogliamo bene all'Italia. Noi vogliamo bene all'Italia, non chi vuole i pieni poteri per farne non si sa che cosa e per andare in ginocchio davanti al governo cinese. Il tutto, Ministro, di fronte a una situazione ben al di sotto di quello che ci state raccontando, perché i contagi comunque sono ben al di sotto della media europea, i contagiati non hanno quella carica virale che tutti temevamo e di conseguenza sappiamo benissimo che i pieni poteri che state cercando servono solamente per togliere le libertà democratiche nel nostro Paese. *(Applausi)*. Questa è l'essenza di questo Governo: togliere le libertà democratiche al nostro Paese, in uno Stato, signor Ministro, dove proprio in vista della stagione turistica si è permesso di tutto e di più, permesso di tutto e di più, senza controlli, perché chi doveva controllare non ha controllato, per poi puntare il dito sulle Regioni, per poi dire che il Presidente della Regione Sardegna è stato inefficiente. Io esprimo la mia solidarietà personale al Presidente della Regione Sardegna. *(Applausi)*. Quando aveva avanzato proposte su come dovevano essere gestiti i turisti in Regione Sardegna l'avete tutti irriso e avete detto che era un irresponsabile; irresponsabile; adesso la colpa è delle discoteche e ci sentiamo dire dai tromboni della politica e da chi fa il fenomeno che la colpa è dei giovani perché non ascoltano, la colpa è dei giovani perché si abbracciano, la colpa è dei giovani perché non mettono le mascherine. Visto che i giovani non mettono le mascherine dovevate prevedere dei controlli e delle sanzioni. Non l'avete fatto e questo è il risultato. Non è colpa dei giovani, è colpa vostra che fate le leggi e non le fate applicare, signor Ministro. In questi mesi, come le abbiamo detto, siamo sempre stati collaborativi. Speravamo che arrivasse qualcosa, perché erano i mesi di calma in cui ci aspettavamo che tutti i tecnici che avete consultato ci dicessero come avremmo dovuto affrontare l'autunno. Noi stiamo affrontando l'autunno facendoci il segno della croce. Sulla sanità. Tornano i turisti dall'estero e dalla Sardegna, Ministro, e non ci sono regole condivise per i tamponi: code chilometriche davanti agli ospedali, giorni per gli esiti dei tamponi e stiamo parlando di qualche decina di migliaia di turisti. Mi immagino se - speriamo di no - dovesse succedere la stessa cosa che è successa questo inverno. Avete avuto il tempo per fare, decidere e condividere con le Regioni e non avete fatto nulla. Sulla scuola mi sembra di sparare sulla Croce Rossa: un Ministro inadeguato, un Ministro che per mesi ci ha raccontato tutto e il contrario di tutto. Fate un rimpasto di Governo e sostituitela. Prima parlava delle distanze, poi parlava dei banchi con le rotelle, poi le mascherine sì, le mascherine no, le mascherine boh; gli orari e i giorni alternati, le scuole e gli spazi da trovare, con 140.000 studenti che devono ancora essere posizionati; il tampone per gli insegnanti sì, il tampone per gli insegnanti no; trasporto degli alunni che è un'odissea. Signori, le cose devono essere chiare. Le famiglie si aspettano risposte chiare. Le famiglie si aspettano di poter mandare i loro figli a scuola nel modo più sereno possibile e di avere un Ministro alla loro altezza. Questo è un Ministro che non è all'altezza delle famiglie italiane.

uno Stato in cui c'è un *Premier* con i pieni poteri deve far rispettare le regole a chi entra irregolarmente nel nostro Paese (perché questi sono irregolari che entrano nel nostro Paese), soprattutto se questi irregolari pensano di fare quello che vogliono. Se entri in modo irregolare nel nostro Paese, stai dove il nostro Paese ti mette, ti piaccia o non ti piaccia. *(Applausi)*. Ministro, siamo molto preoccupati. Informazioni tenute nascoste ai cittadini, con metodologie da ex Unione Sovietica; pieni poteri a un *Premier* con limitazione delle libertà previste dalla Costituzione; confusione e mancanza di programmazione dei servizi fondamentali previsti dalla Costituzione (istruzione e sanità).

che il senatore Monti, quando era *Premier*, è stato quello che ha tagliato la sanità in Italia? *(Applausi)*. In un momento di crisi mondiale, all'Organizzazione mondiale della sanità noi mettiamo quello che ha massacrato la sanità nel nostro Paese. Siamo la repubblica delle banane, se abbiamo solamente il senatore Monti all'Organizzazione mondiale della sanità. Bastava prendere uno di quelli che voi chiamate eroi e mandarlo all'Organizzazione mondiale della sanità. Perché quelli non sono eroi solamente in Aula: bisogna riconoscere il loro lavoro anche dando loro ciò che meritano.

l'interessante, rigorosa e seria, come sempre, relazione del ministro Speranza, rispetto alle priorità che in un Paese normale sarebbero condivise:

nel pieno di una pandemia, in cui abbiamo ancora di fronte mesi difficili e in cui dobbiamo con fatica riuscire a far convivere due cose, che naturalmente non convivono. la relazione e la socialità non convivono con la prevenzione da un virus che si trasmette esattamente attraverso la relazione e la socialità. Abbiamo attraversato mesi drammatici, in cui abbiamo dovuto dovuto interrompere drasticamente la relazione e la socialità; abbiamo accettato la sfida, tutti insieme, maggioranza e Governo, di provare a vivere la relazione e la socialità socialità in sicurezza. È una grande sfida, che comporta un rafforzamento dei nostri sistemi sanitari, come il Ministro ha spiegato in maniera molto chiara, una tempestività nell'intervento, una capacità di reazione, una capacità di presenza sul territorio. Ma comporta anche un'indicazione dei comportamenti da seguire da parte delle persone che non si limiti agli aspetti tecnici. Non si tratta solo di imparare, quando governi la nave, come si alzano le vele; si tratta anche di capire in che direzione andare, come interpretare le stelle. Questo è uno dei compiti della politica. Un Paese si comporta anche secondo la classe dirigente che ha, la classe dirigente di questo Paese si deve assumere la responsabilità di mandare dei messaggi ai propri cittadini sui comportamenti da avere nei prossimi mesi. Sarebbe stato utile anche negli ultimi mesi, perché noi avremmo potuto, durante l'estate, arrivare a contagio zero, se non ci fossero stati alcuni comportamenti scellerati, di cui non sono responsabili, come qualcuno dice che noi diciamo - e non lo diciamo mai -, ad esempio i nostri ragazzi, però certi pifferai magici sì, certi Lucignolo che portano i ragazzi nei paesi dei balocchi sì: loro sono responsabili, perché quest'estate non era il momento di abbassare i comportamenti di cautela. Allora ci sono dei responsabili. Io mi occupo di spettacolo dal vivo ed ho un grande rispetto per il *cabaret*, che è una grande arte. Ma non mi aspettavo oggi di sentire in quest'Aula delle forme di *cabaret* *(Applausi),* perché in questi mesi non c'è proprio niente su cui scherzare; proprio niente su cui scherzare; non c'è da fare le battute, come alle scuole medie, sui cognomi dei colleghi in un momento di pandemia persone in quest'Aula che hanno una storia politica ben più lunga della mia, che siedono in questi banchi da numerose decine di anni, che dovrebbero aver maturato la serietà di comportamento, la serietà di comportarsi in maniera responsabile in un momento in cui si scherza con la vita delle persone. Allora finiamola finiamola di inventarci dei nemici che non ci sono. Nel bellissimo ultimo film della saga sull'Uomo ragno c'è un signore che non è un supereroe ma che ha costruito dei cattivi immaginari che si vedono grazie a dei proiettori; lui li sconfigge e diventa un supereroe. Noi in quest'Aula continuiamo a vedere qualcuno che vuole fare il supereroe, sconfiggere dei nemici che non ci sono, che stanno per invadere questo Paese ogni mezzo minuto, quando invece c'è un nemico vero, microscopico, invisibile, che dobbiamo sconfiggere tutti insieme e che richiede un salto di qualità e di responsabilità da parte di tutti. Signor Ministro, guardi io la ringrazio non solo per il lavoro straordinario che ha fatto in questi mesi, ma anche per il suo rigore, per il suo comportamento e per il suo atteggiamento. Noi - e non è piaggeria questa, perché ci conosciamo da tanti anni e non abbiamo bisogno di fare queste cose - abbiamo bisogno di politici che abbiano questo tipo di comportamento e di atteggiamento,

abbiamo bisogno di un campo conservatore come di un campo progressista. Però abbiamo bisogno di *leader* conservatori, che si dividono con noi su tanti provvedimenti e su quali sono le strategie di fondo dell'economia, ma che non si dividono quando c'è da affrontare insieme una pandemia. Anche io non ho piacere a stare nella stessa barca con alcune persone, però in questa barca ci siamo e allora dobbiamo provare tutti a remare nella stessa direzione, altrimenti veniamo mangiati dai coccodrilli. Ci piaccia o meno. Quando sei naufrago sull'isola deserta ti fai andare bene anche il collega che hai. Quindi facciamo tutti uno sforzo. Non ci vorremo sicuramente bene, però almeno proviamo ad arrivare al vaccino senza utilizzare per la campagna elettorale tutte le armi disponibili, assolutamente disinteressandoci del futuro dei nostri ragazzi, dei nostri bambini e dei nostri anziani, che rischiano la vita nei prossimi mesi. Non sono un allarmista però questo è un dato di realtà. Voglio Voglio parlare al cuore, ma voglio anche fare un monito: guardate, non metteteci nella condizione tra qualche mese di dovervi dire che siete responsabili delle persone che torneremo forse a perdere, perché c'è l'emergenza oppure no. Non ci sarà Non ci sarà l'emergenza oggi nelle sale di terapia intensiva, ma non c'è per le cose drammatiche che abbiamo dovuto fare nei mesi scorsi. Vogliamo tornare a quelle cose drammatiche? Vogliamo tornare all'emergenza nelle sale di terapia intensiva o vogliamo dire che la pandemia fino a che non c'è un vaccino è un'emergenza e che non se l'inventa nessuno? *(Applausi).* Come si fa a dire che qualcuno vuole limitare le libertà? Chi è al Governo, se avesse la possibilità, direbbe ai suoi cittadini, anche per opportunismo, di divertirsi e di fare tutto quello che ritengono, ma purtroppo questo non lo possiamo fare e quindi facciamo un salto di qualità nella cultura e nella qualità della classe dirigente, che affronti la

PIRRO *(M5S)*. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, parrebbe che improvvisamente qualcuno si sia reso conto che il virus Sars-Cov-2 è ancora in circolazione e fa paura. Ora tutti paventano una seconda ondata, magari dopo aver avuto comportamenti imprudenti. I dati delle ultime settimane confermano che era necessario prorogare lo stato di emergenza, come ci eravamo detti in questa stessa Aula poco più di un mese fa. Ancora una volta, grazie alle scelte coraggiose e responsabili di questo Governo, elogiate dalla comunità scientifica mondiale, abbiamo tenuto a bada i contagi, contrariamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei, che dopo una prima ondata apparentemente più modesta che in Italia ora si trovano ad affrontare numeri di contagi giornalieri molto alti. In questi mesi abbiamo messo in atto misure e strategie di intervento tali da mettere in sicurezza il nostro Servizio sanitario nazionale, come ad esempio l'effettuazione di tamponi a chi rientra da zone ad alto rischio, anche col sistema del *pit stop* e senza le code che qualcuno ha immaginato (lunedì ero in un ospedale, c'era il servizio di *pit stop* e non c'era nessuna attesa per effettuare il tampone). Stiamo incrementando sempre di più il numero dei tamponi che effettuiamo giornalmente, che vanno ancora aumentati in vista della riapertura delle scuole ed oggi abbiamo superato il numero di 100.000. Questo ci consente di individuare tutti quegli asintomatici che a marzo e ad aprile ci sfuggivano, perché contrariamente a quanto ha affermato ad esempio il senatore Zaffini, non ci limitiamo più a testare solo chi manifesta i sintomi, ma tracciamo più accuratamente la catena dei contagi e i comportamenti a rischio. Questo è fondamentale per circoscrivere i focolai e consentirci di guardare con serenità al prossimo importante appuntamento, che è la riapertura delle scuole, perché questa è la nostra priorità assoluta, come ha giustamente detto anche lei, signor Ministro. Ogni nostro sforzo e ogni sacrificio mirano a questo risultato. Dovremmo mettere fine alle polemiche. Avremmo dovuto lavorare tutti insieme con questo obiettivo in maniera trasversale e invece così non è stato, si e colta l'occasione per attaccare il ministro Azzolina, a cui vanno tutto il nostro appoggio e la nostra solidarietà non solo perché sta facendo un ottimo lavoro e sta risolvendo problemi causati anche da decenni di cattiva amministrazione della scuola, ma anche e soprattutto per i beceri attacchi sessisti che riceve continuamente, in particolare sulle pagine dei simpatizzanti di un certo partito. Purtroppo accade troppo spesso che chi si sente inferiore non abbia strumenti per controbattere e non trovi di meglio da dire che qualche frase offensiva, che non avendo grandi strumenti intellettivi basi il proprio modo di ragionare sulla propria mascolinità e non riesca ad accettare di soccombere dinanzi ad una giovane donna preparata ed anche bella. *(Applausi)*. Ma se ne facciano una ragione: Lucia è migliore di loro, migliore di chi abbandona la barca quanto teme che stia affondando. Per fortuna c'è chi non fugge dinanzi ai problemi e riporta la barca in porto sana e salva. Colgo l'occasione per rispondere anche ad un'altra sciocca affermazione dell'ex Ministro leghista, che non accettava lezioni da chi parla di scie chimiche. Ebbene, siamo noi che non vogliamo stare sulla stessa barca di chi siede vicino e milita nel partito di chi nel luglio del 2013 presentò un'interrogazione al Parlamento europeo proprio sulle scie chimiche e la loro pericolosità. Ma torniamo ad oggi. Dovremmo tutti insieme responsabilizzare i nostri figli, i nostri giovani al rispetto delle tre semplici regole ritenute fondamentali dalla comunità scientifica mondiale: indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani, mantenere le distanze. Smettiamola di parlare di banchi con le rotelle. Ormai è evidente a tutti che questi sono solo una minima parte di quelli ordinati e saranno utilizzati per forme di didattica finalmente più moderna e alternativa a quella tradizionale. Poniamo invece attenzione affinché gli enti territoriali mettano correttamente in pratica le linee guida sul trasporto pubblico locale, cosicché i nostri ragazzi possano arrivare a scuola in totale sicurezza. Questi sono gli aspetti fondamentali in questo momento: la sicurezza sanitaria del Paese, non abbassare la guardia e fare ogni sforzo perché la ripresa in corso sia delle nostre attività sociali, che del tessuto economico non sia messa a rischio, ma - anzi - supportata, sostenuta e agevolata. Queste dovrebbero essere le priorità di tutti e non misere polemiche sterili e vergognose da campagna elettorale. Vigiliamo piuttosto insieme affinché le Regioni presentino velocemente i piani per la riduzione delle liste d'attesa e per l'utilizzo dei quasi 500 milioni di euro messi a disposizione con il cosiddetto visto che siamo tutti concordi nel ritenere una criticità il fatto che, a causa del *lockdown*, molti cittadini non hanno trovato risposta alle loro necessità e che ora bisogna rimediare. Dimostriamo di essere responsabili e pensiamo al bene dei nostri concittadini. Noi lo siamo e lo saremo sempre e per questo annuncio convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione della maggioranza.

Signor Presidente, signor Ministro, ho sentito con sincero dispiacere dai banchi dell'opposizione apostrofare il Governo con parole tipo «criminali». Penso che il Governo abbia agito sostanzialmente bene nel periodo di effettiva emergenza e condivido anche quanto detto dal ministro Speranza sul fatto che occorre mantenere prudenza. Tuttavia, non penso che la prudenza sia incompatibile con gli strumenti ordinari

tra gli impegni del Governo, quello di revocare lo stato di emergenza, che invece è stato prorogato al 15 ottobre. Mi aspettavo ciò specie leggendo nelle premesse della proposta di risoluzione di maggioranza quanto segue: «Dai dati epidemiologici risulta complessivamente che il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Covid-19 in Italia non manifesta particolari criticità». Date queste premesse, mi sarei aspettato la richiesta al Governo di revocare lo stato di emergenza, così come che ci fosse una richiesta all'Esecutivo di massima trasparenza e di pubblicizzare tutti gli atti del Comitato tecnico-scientifico. Questa colpevole omissione presente nella proposta di risoluzione ha consentito a personaggi tra i più politicamente torbidi e opachi della storia del del nostro Paese, come il senatore Gasparri, di fare a noi del MoVimento 5 Stelle una lezione sulla trasparenza. Pertanto, date queste colpevoli omissioni,

relativamente all'attuale riacutizzarsi del contagio da coronavirus mi permetto di rammentarle che già nel mese di febbraio scorso ho ritenuto opportuno suggerire il ricorso alle proprietà terapeutiche derivanti dagli estratti di *cannabis* al fine di contrastare... *(Commenti).* Presidente, io ho bisogno di parlare.

e, quantomeno inizialmente, non si è potuto neanche accertare l'esatto decorso della patologia viste le mancate autopsie. Solo per l'intervento di alcuni medici più coraggiosi, sebbene in un momento successivo, si è potuto accertare che le infiammazioni diffuse e le tempeste citochiniche indotte dal virus sono causa di trombosi che paralizzano l'apparato cardiorespiratorio sino a indurre il decesso. Ebbene, è notizia già di alcuni mesi fa che l'utilizzo degli estratti di cannabis può concretamente combattere gli effetti del Covid-19. Il Medical college of Georgia ha infatti pubblicato sulla rivista scientifica «Cannabis and cannabinoid research» i risultati di uno studio, concludendo che il CBD potrebbe aiutare chi si ammala in modo grave di Covid. Non ritengo, Ministro, che si possa ignorare consapevolmente l'esistenza di valide alternative a un vaccino non ancora reso disponibile né tantomeno ritengo condivisibile limitarsi a prorogare le attuali misure di contenimento senza valutare adeguatamente l'adozione di una terapia risolutiva o quantomeno coadiuvante nella lotta al virus. mi vedo quindi costretto a esternare il mio voto contrario a un'ulteriore inoperosa attesa della produzione di un possibile vaccino farmacologico con proroga delle attuali misure di contenimento che si sono rilevate limitatamente efficaci, e ciò ove si consideri che quantomeno nel frattempo si può far ricorso a una terapia alternativa, priva peraltro di effetti collaterali noti. PRESIDENTE.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

evitiamo gli assembramenti. Se volete, uscite in maniera ordinata in modo che il senatore Bossi possa iniziare il proprio intervento. Prego, senatore.

Signor Presidente, di solito negli interventi di fine seduta riportiamo notizie tragiche e talvolta drammatiche, mentre stavolta vorrei andare controcorrente e portare l'Assemblea a conoscenza di una buona notizia. Nella mattinata del 23 agosto, peraltro giorno del mio compleanno - e la ringrazio per gli auguri che mi ha fatto pervenire - nel delta del Po e più precisamente nei Comuni di Taglio di Po e Goro, il personale del Gruppo dei Carabinieri forestali di Rovigo e delle stazioni dipendenti - vorrei citarli uno a uno, ma per mancanza di tempo citerei solo coloro che si sono distinti in modo particolare: il tenente colonnello Alessandro De Vido e il maresciallo Stefano Zanghierato, del Gruppo carabinieri forestali di Rovigo, mentre per la Soarda, la sezione operativa antibracconaggio reati a danno degli animali, il maggiore Testa e il brigadiere capo Rossano Tozzi - coordinati dal pubblico nell'operazione denominata Gold River - hanno sgominato una vera e propria banda di pescatori di frodo, i famosi bracconieri. Secondo le contestazioni notificate, questo gruppo era uno dei più importanti cartelli di predoni delle aste fluviali, che spaziavano in tutta Italia, un vero e proprio quartier generale della commercializzazione illecita del pescato catturato per poi essere rivenduto al mercato estero, in violazione delle norme vigenti e in modo non conforme alle normative sanitarie, mascherata dietro l'attività professionale di alcuni di loro. 16 le persone di nazionalità rumena e una ungherese indagate, più di 50 persone sono coinvolte nella rete per aspetti amministrativi, immobili e veicoli sono stati sequestrati e ad otto di questi individui è stata infine contestata l'associazione per delinquere.

nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid hanno continuato a lavorare e a verificare con determinazione quanto è emerso ancora una volta. volta. Mi riferisco a ciò che io ed altri colleghi abbiamo portato all'attenzione pubblica e delle istituzioni. Abbiamo votato in questo ramo del Parlamento, nell'arco di tre mesi, in sede deliberante - dando la dimostrazione al Paese intero che, se si vuole, le cose si possono fare - una legge per permettere di fermare reati di questo tipo. Purtroppo questa proposta di legge, signor Presidente, è ancora ferma alla Camera del Parlamento non hanno la nostra sensibilità, oppure fanno finta di non averla. Questa proposta di legge è calendarizzata in Commissione agricoltura e aspetta solo di essere licenziata: un lavoro volenteroso, che volendo si fa in due settimane.

ricordo che queste bande criminali il più delle volte sono armate e pericolose e ricordo che dietro le divise dei volontari che controllano i fiumi ci potrebbero essere i vostri figli e i vostri mariti. Quindi non aspettiamo che ci scappi il morto, per rendere realtà questa

delle professioni sanitarie, che è previsto come strumento di collegamento tra il Ministero dell'università e il Ministero della salute, perché ha precisamente come obiettivo specifico quello di verificare la programmazione del numero di posti da mettere a concorso nei diversi corsi di laurea

(medici, infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio) è massima, abbiamo dimenticato totalmente di prestare l'attenzione dovuta a coloro che per legge sono preposti a prendere decisioni, come uno di quei (chiamiamoli così) previsti come organi di consultazione dei rispettivi Ministri, ma anche come organi di collegamento con i collegi professionali. Io chiedo quindi che il rinnovo dell'Osservatorio delle professioni sanitarie trovi l'attenzione dovuta sia per l'emergenza che stiamo vivendo, sia per il rispetto ordinario a professionalità di alta qualità a cui è affidata la salute di tutti noi, nella doppia prospettiva diagnostica, come succede per alcuni di questi profili (penso ai tecnici di radiologia e di laboratorio), e terapeutica, come succede ad altri di questi profili professionali (fisioterapisti, logoterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva e così via). In questo momento, totalmente attenti e totalmente fagocitati dall'emergenza Covid, stiamo dimenticando tutto il resto della sanità, stiamo dimenticando di rendere non un omaggio, ma la dovuta attenzione a coloro che di fatto si prodigano in tutti gli ambiti della sanità. sanità. Credo sia importante che concretamente il Ministro dell'università e il Ministro della salute, con un'azione coordinata e combinata, ridiano spazio all'Osservatorio delle professioni sanitarie. Lo attendono centinaia di migliaia di professionisti; oltre 400.000 professionisti, tra infermieri e tutti gli altri, stanno aspettando di vedere riconosciuta... Grazie

del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso